restringe il livello di concorrenza e consente alle autorità pubbliche, alle amministrazioni e alle stazioni appaltanti di evitare le gare,

Non sto a citare le norme, ma è estremamente evidente che elevare da 500.000 ad un milione di euro il limite di importo entro il quale è consentito affidare i lavori con la procedura negoziata senza bando, anche per i beni culturali, significa non andare nella direzione che voi stessi avete indicato. Voglio ricordare - l'ho qui con me il disegno di legge n. 2156, presentato dal Ministro della giustizia, che reca «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione».

lo stesso Governo e la stessa maggioranza propongono delle norme assolutamente contrarie a quelle contenute nell'articolo 4 di cui sto parlando. Del resto, la stessa contraddizione la troviamo con il Piano casa.

Per non parlare del credito d'imposta, che sicuramente è un fatto positivo, ma che avete limitato ad una parte incrementale, e non a ciò che invece le aziende realmente possono spendere o hanno speso per la ricerca. l'ennesima fiducia con cui ci accingiamo ad approvare questo decreto impedisce una vita parlamentare costruttiva. Questa fretta continua è intervallata da pause in cui il Senato produce soltanto mozioni e ordini del giorno, cioè nulla, sul piano dell'azione dell'azione legislativa. Quando si tratta di affrontare temi seri e importanti, lavoriamo con la fretta determinata dalla scadenza dei decreti, e questo impedisce che il Parlamento possa dare un contributo. Ad esempio, noi abbiamo presentato degli emendamenti che aiutavano il Governo a poter subito realizzare il credito d'imposta, senza attendere l'autorizzazione europea, sfruttando anche le risorse FAS per 11 miliardi: tutto questo non è possibile. Ci troviamo come sempre davanti a un muro. Il Governo sta lì ad ascoltare passivamente - altrimenti la seduta non è valida - e l'opposizione è costretta ad esprimere le proprie proposte, a rappresentarle, ma in un dialogo senza vita, senz'anima. Questa è la ragione più profonda del dissenso nei confronti del merito della fiducia. Voi del resto la rimetterete sicuramente anche sulla manovra finanziaria. È un modo di dire: è inutile che il come del resto qualcuno non ha mancato di affermare in altre occasioni. E poi l'articolo 9 sulla scuola: è un articolo che dovrebbe diffondere qualche speranza soprattutto nel mondo dei precari, ma che a ben leggere sega queste speranze. Anzitutto, quanto alla nuova idea della Fondazione per il merito, chiedo al Sottosegretario: in un Paese in cui si invoca da più parti la semplificazione si vuole evitare assolutamente di mettere su nuovi carrozzoni, per poter organizzare il Fondo per il merito previsto dalla legge n. 240 del 2010, istituiamo un'altra Fondazione

la cancellazione di quella norma che prevede la riserva della quota del 10 per cento per gli studenti iscritti all'università che sono residenti in quella Regione; una norma, a mio avviso, assolutamente anticostituzionale e discriminante, che non aiuta a valutare ed incentivare il vero merito. Abbiamo portato proposte anche in ordine al dramma dei pagamenti ritardati per le imprese, ma non ho il tempo di affrontare questo tema. Voglio concludere dicendo che la vita parlamentare soffre terribilmente, e quindi il Paese, il bene comune del Paese soffre di questa voluta mancanza di dialogo. Noi avevamo, sempre nell'invarianza dei saldi di bilancio, fatto proposte che avrebbero sicuramente migliorato questo testo; invece, ci troviamo a dover scegliere ineluttabilmente la strada della parola,

onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire si inserisce nell'ambito delle indicazioni e delle misure economiche stabilite da Bruxelles per il semestre europeo: misure estremamente importanti e indispensabili, che ci permettono di condividere non soltanto la dimensione europea del nostro Paese, ma anche le politiche economiche dettate dall'Unione europea. decisioni improcrastinabili di fronte alle possibili speculazioni finanziarie internazionali che interesserebbero il nostro Paese qualora non fosse in grado di assumere scelte e interventi che sostengono il mondo delle imprese e le famiglie. È importante contestualizzare, soprattutto per la delicatezza della materia che oggi affrontiamo con grande responsabilità, gli effetti devastanti che la crisi economico-finanziaria sta producendo a pochi chilometri da noi. Le immagini che quotidianamente ci arrivano dal subbuglio delle piazze greche devono far riflettere chi oggi si assume la responsabilità di non voler concorrere a sostenere, esercitando democraticamente il ruolo dell'opposizione, proposte migliorative di provvedimenti in favore di tutte le aree che producono sviluppo nel nostro Paese, da chi produce ricchezza a chi produce consumo. decreto sviluppo sono inserite disposizioni di contrasto alla crisi finanziaria e alla crisi dei mercati oltre a norme a favore dell'economia reale e del mondo delle imprese. In primo luogo, il provvedimento costituisce un contributo positivo all'economia italiana e al rilancio del mondo del lavoro rispetto alle tante riforme fatte in vari ambiti dell'economia

Le aree relative ai distretti turistici saranno a «burocrazia zero»: mi preme quindi sottolineare anche come questa norma rilancerà gli investimenti del settore turistico-balneare, fondamentale nel nostro Paese. I contingentati tempi per 1'approvazione da parte del Senato di questo decreto, causati anche dall'importantissima manovra finanziaria che il nostro Parlamento attende per 1'approvazione, non ci consentono tuttavia ulteriori approfondimenti rispetto ad un testo che è comunque fonte di sviluppo per i tanti settori della produzione e del consumo. Norma rilevante è quella che prevede l'impossibilità di apporre ipoteche sulla prima casa per crediti fiscali inferiori ai 20.000 euro, analogamente a quanto disposto per gli espropri. Il cosiddetto decreto sviluppo facilita e semplifica le procedure di rilascio dei documenti di identificazione dei cittadini prevedendo, tra 1'altro, 1'unificazione, anche progressiva, della carta di identità elettronica con la tessera sanitaria. Con il decreto che approveremo, torna ai Comuni la funzione della riscossione delle entrate precedentemente affidata ad Equitalia, allentando la presa, forse eccessiva, sui contribuenti. Norma in favore delle famiglie è quella sui mutui casa: ovvero si consente con questo decreto 1'ampliamento della platea dei destinatari della disciplina sulla rinegoziazione dei mutui ipotecari a tasso variabile. L'Italia ha bisogno di uscire da questa situazione con una politica seria e rigorosa. Questo decreto costituirà un contributo positivo per l'economia italiana e per il rilancio del mondo del lavoro rispetto alle tante riforme fatte in ambiti vari - come prima dicevo - dell'economia. un rilancio responsabile che passa attraverso 1'assunzione di provvedimenti, come questo che non avrà sostanzialmente alcun impatto sui conti pubblici, così come certificato dalla Relazione tecnica «bollinata» dalla Ragioneria dello Stato, e che quindi non comporta ulteriori effetti negativi sulla spesa. Per questo motivo, oltre agli elementi positivi evidenziati nel mio intervento, il Gruppo di Coesione Nazionale-Io Sud garantisce, anche con autonomia propositiva, il proprio sostegno a tutte quelle misure che vorranno evitare all'Italia una fase di incertezza e di instabilità;

insieme contemporaneamente il federalismo fiscale e la delega sulla perequazione infrastrutturale. Il federalismo, infatti, può tenere insieme questo Paese, può renderlo più competitivo e responsabile, ma guardandosi gli uni con gli altri senza reciproche demonizzazioni, perché la capacità da ricercare non è quella di rompere, ma quella di unire, di condividere,

Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame si colloca in una congiuntura economica particolarmente difficile per l'intera Europa. L'Italia, al pari dei Paesi più esposti alle pressioni della finanza internazionale che ha scombussolato il mercato, ha dovuto affrontare una crisi economica di sistema che l'ha costretta ad una forte azione di rigore dei conti economici. La preoccupazione, che è stata ed è ancora viva, è di riuscire a contenere l'indebitamento, da coniugare con un sostegno alle fasce più deboli, e contestualmente di mettere in campo alcune misure atte a favorire la crescita, quest'ultima vera garanzia non solo per una ripresa economica, ma per una sostenibile tenuta dei conti pubblici. Le disposizioni in esame si propongono questo obiettivo che, oggi, alla luce della manovra economica varata dal Consiglio dei ministri giovedì della scorsa settimana, assume un valore da derubricare a provvedimenti acquisiti. È tuttavia importante in questa fase del dibattito parlamentare ricordare e fotografare quanto di buono è contenuto nella norma, ma anche le difficoltà e le discutibili scelte che, se corrette, possono effettivamente traghettare, con l'aiuto della prossima manovra economica, la nostra Nazione fuori dalla palude confusa della crisi, secondo le indicazioni della Comunità europea. Per ragioni di spazio e di tempo mi atterrò alle sole questioni relative agli interventi infrastrutturali ed alle semplificazioni urbanistiche.

negli strumenti attuativi le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia sono eseguite direttamente dal titolare del permesso di costruire; sono eliminate le procedure negoziate del codice degli appalti; è introdotto il silenzio assenso per il rilascio del permesso di costruire; è permessa la tolleranza del 2 per singola unità immobiliare per le lievi difformità relative ad altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta: è introdotta la SCIA in edilizia, che non sostituisce la super super DIA; sono previste semplificazioni burocratiche e temporali, ad esempio per le costruzioni (la SCIA può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento e vale la data di ricevimento); i diritti edificatori sono ricompresi nell'ambito dei diritti reali; i relativi contratti di trasferimento sono soggetti a trascrizione nei registri immobiliari. Molto positivi sono gli interventi sulla VAS, così come le disposizioni in tema di riqualificazione delle aree urbane degradate,

agli interventi di riqualificazione del permesso di costruire in deroga anche per il mutamento di destinazione d'uso; l'ammissibilità in via generale del rilascio del permesso di costruire in deroga anche per il mutamento di destinazione d'uso, purché compatibile o complementare; l'approvazione in via generale

In realtà, noi avremmo preferito veder discusso e approvato il disegno di legge di cui sono primo firmatario insieme ai colleghi senatori Piscitelli e Villari del Gruppo di Coesione Nazionale-Io Sud, contenente disposizioni in materia di rigenerazione urbana per favorire la capacità abitativa e l'incremento delle aree verdi. Questo disegno di legge può veramente contribuire a cambiare in modo qualificato il sistema residenziale tanto dal punto di vista abitativo quanto sotto il profilo ambientale e ciò con particolare riferimento alle grandi periferie urbane. Sul versante infrastrutturale ricorre l'obbligo di ricordare alcuni dati. In Italia permane una situazione di forte crisi che, secondo le valutazione dell'ANCE, non si è esaurita nel 2010 ma prosegue anche quest'anno e nel prossimo 2012.

Nel 2011 l'ANCE rileva un peggioramento delle aspettative produttive rispetto alle attese manifestate dalle imprese nel settembre scorso, che si concretizza con una flessione degli investimenti in costruzioni, previsti del 4 per cento, contro la precedente indicazione del 2,4 In assenza di misure che possano introdurre effetti immediati sulla produzione (che purtroppo in questo decreto non ci sono), anche per il 2012 si prospetta una ulteriore riduzione del 3,2 In 4 anni, dal 2008 al 2011, il settore delle costruzioni avrà perso il 19,8 per cento in termini di investimenti. La produzione di nuove abitazioni si è ridotta del 35,5 per cento, l'edilizia non residenziale privata è diminuita del 19,2 I lavori pubblici, nello stesso periodo, sono diminuiti del 28,7 per cento, ma, se si tiene conto dell'andamento negativo già in atto dal 2005, il calo produttivo raggiunge il 34,8 Con riferimento all'occupazione dipendente e considerando che il calo delle ore lavorate è di circa il 19 per cento dall'inizio della crisi, si stima che i posti di lavoro persi nelle costruzioni siano circa 230.000; considerando anche gli effetti sui collegati, la perdita di occupazione sale così a circa 350.000 unità. D'altra parte, nonostante l'Italia abbia un'incidenza della spesa pubblica corrente e in conto capitale sul PIL tra le più elevate d'Europa (52,5 per destina agli investimenti fissi lordi solo una parte modesta della spesa (2,5 per cento del PIL). Quest'ultimo dato, riferito al 2009, risulta ancora più basso per il 2010 (2,1 per cento) e diminuirà ancora probabilmente quest'anno. Appare troppo evidente la necessità di abbattere il debito contraendo la cassa, ma l'effetto è quello che abbiamo appena descritto. Ciò significa percorrere sempre di più la strada del rigore dei conti che, in questo caso, si oppone però a quella della crescita. Il provvedimento non incide pertanto, purtroppo, a nostro modesto avviso, sui meccanismi della crescita, anche se dobbiamo apprezzare lo sforzo che è stato fatto per favorire, così come previsto all'articolo 4, modifiche importanti in materia di contratti pubblici e, in particolare, al codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Le modifiche sono finalizzate a ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, a semplificare le procedure di affidamento, a garantire un più efficace controllo e a ridurre il contenzioso. Un ultimo capitolo che ci pare meritasse di essere considerato in un decreto che si pone come obiettivo lo sviluppo del Paese è quello della liberalizzazione del sistema. Così come ricorda l'Autorità per la vigilanza sui contratti di lavoro, servizi e forniture nella sua Relazione annuale del 2010, nel paragrafo «segnalazioni al Parlamento», la qualità dell'allocazione delle risorse pubbliche dipende soprattutto dal livello di trasparenza del procedimento amministrativo e dall'effettiva concorrenza tra gli operatori economici coinvolti. L'Autorità ha pertanto ritenuto opportuno segnalare alcuni interventi volti a rimuovere ostacoli alla concorrenza. In particolare, è emerso un notevole incremento del ricorso alla procedura negoziata senza bando di gara anche a seguito dell'innalzamento della soglia per i lavori pubblici a 500.000 euro. Al fine di limitare tale pratica anticoncorrenziale - dice l'Autorità - sarebbe stata opportuna una modifica normativa volta a porre un termine temporale alla citata disposizione, integrando la stessa con il riferimento al principio dell'adeguata pubblicità e all'elenco per l'individuazione dei soggetti da invitare. Per quanto riguarda i concessionari di lavori pubblici, occorre un maggiore controllo sul rispetto di affidare a terzi una quota di lavori a tutela della concorrenza. Sarebbe stato auspicabile pertanto un incremento, già in questo decreto, della quota da affidare a terzi ben superiore al 30 per cento e l'introduzione dell'obbligo per il concessionario di documentare i lavori di appalto a terzi con cadenza periodica, secondo piani prestabiliti dalle parti. Secondo l'Autorità e secondo il nostro modesto parere, si pone anche una sorta di riqualificazione delle stazioni appaltanti e, a giudizio di chi parla, anche delle SOA. Purtroppo ciò non è contenuto nell'attuale decreto, né esistono norme per favorire o diminuire - come detto - le quote dei lavori *in house* e la relativa possibilità di aprire il mercato alla oggi carente offerta per le progettazioni o i servizi di ingegneria in generale. Si pensi che le gare di ingegneria e architettura, non solo infrastrutturali, nel primo quadrimestre del 2011 sono ai minimi storici: appena 1.446, per un valore di 168 milioni di euro,

Signora Presidente, onorevoli colleghi, in conclusione io credo che si possa accettare questo decreto come un segnale positivo e di disponibilità dell'Esecutivo, anche anche se gli aspetti che ho trattato meritavano di essere allocati in provvedimenti organici che potessero avere una continuità di esistenza normativa coerente con la liberalizzazione del mercato europeo e fossero improntati alla crescita.

finalmente una notizia positiva per il nostro Paese, specie dopo che per tre anni il Governo e questa maggioranza hanno cancellato in generale il tema del governo dell'economia in una fase di crisi che non ha precedenti da oltre 90 anni.

limitandosi viceversa - unico Governo al mondo - a un puro galleggiamento, con risultati drammatici per le imprese e la loro capacità di reggere la nuova competizione internazionale, per i lavoratori, per l'occupazione, le donne, i giovani, per i precari che hanno pagato per primi e di più gli effetti della crisi stessa e poi per i redditi, per quel vero e proprio processo di impoverimento che ha creato una debolezza assoluta della domanda interna, determinando un problema assai serio ai fini della crescita e dello sviluppo. Quindi, un decreto sullo sviluppo con misure rilevanti e mirate - seppur tardivo e di molto - sarebbe comunque uno strumento assai importante ed una vera e propria notizia per il Paese, anche perché propagandisticamente vi è stato costruito sopra un pezzo non secondario della recente campagna elettorale. Invece si parla di decreto sullo sviluppo quando in realtà ci troviamo davanti a un provvedimento in cui ancora una volta di misure per lo sviluppo e la ripresa economica del Paese non vi è traccia davvero visibile e, soprattutto, all'altezza dell'altisonante denominazione del decreto stesso - il senatore Agostini lo ha spiegato in dettaglio, in modo assolutamente eccellente, cosa che facciamo anche con i nostri mirati emendamenti a meno che il Governo non intenda dare alla parola "sviluppo" un significato del tutto proprio. Allora, non ci resta che ricorrere al dizionario della nostra lingua, cosa sempre utile in questi casi. Esso definisce lo sviluppo economico come «la situazione di un Paese in cui si registra una crescita nel tempo delle principali grandezze economiche (prodotto lordo-netto, investimenti, occupazione, reddito *procapite*), alla quale si accompagna una continua innovazione nelle tecnologie impiegate nella produzione di beni e servizi». Ecco, onorevoli colleghi, se questo è il significato letterale della parola "sviluppo", mi sembra incontrovertibile sostenere che a tale scopo le misure del decreto che esaminiamo siano a dire poco insufficienti (e sto usando, credetemi, parole molto misurate). Quel che è certo, infatti, è che questo decreto non attrezza il Paese a uscire dalla crisi con investimenti mirati o aiuti alle imprese, per non parlare di una politica industriale degna di questo nome (per inciso,

dei redditi da lavoro e da pensione, né tanto meno investimenti in settori come la ricerca, l'innovazione e l'istruzione che costituiscono, come è noto, *asset* strategici dai quali le economie degli altri Paesi nostri competitori sono ripartite nel pieno della crisi e che oggi le fanno più forti: per noi non costituiscono invece le priorità per ridare competitività a tutto il sistema. Allora, ripeto: che significa la parola "sviluppo" per questa maggioranza? Forse la spiegazione è quella rappresentata dall'atteggiamento del Presidente del Consiglio che, presentando la prossima manovra con il Ministro dell'economia e delle finanze, si è detto molto dispiaciuto per la tassa sui SUV, mentre non ha speso neppure una parola per la scure che si sta abbattendo sui pensionati. Eppure, stiamo parlando di un taglio che darà un ulteriore colpo ai redditi di operai e impiegati in pensione, colpendo così, tra l'altro, proprio quella classe media che dite a parole di voler tutelare. La verità è che questo Governo non ha idea di come rimettere in moto il Paese e questo decreto-legge ne è un'ennesima testimonianza. I numeri della crisi non mentono, onorevoli colleghi, e mai come in questo caso parlano da soli, e ci raccontano, in particolare, di categorie sociali meno tutelate: penso alle donne, colpite da un tasso di disoccupazione che arriva al 46 per cento nel Sud e ai giovani, la risorsa più preziosa per il presente e per l'avvenire del nostro Paese. Il tasso di disoccupazione dei giovani sfiora il 30 per cento e ci sono 2 milioni di giovani cosiddetti NEET che sono talmente sfiduciati che neppure più lo cercano, il lavoro. ci parlano anche di chi ha la fortuna di trovarne uno di lavoro e non se la passa certo un granché meglio, perché rimane invischiato nella trappola della precarietà precarietà che impedisce ai nostri ragazzi di decidere liberamente del loro futuro perseguendo le proprie aspirazioni. Ma come si fa a non occuparsi seriamente, in questo che chiamate decreto per lo sviluppo, del tema del lavoro e, in particolare, del precariato? E che senso ha il colpo di mano della ministra Gelmini che all'ultimo momento ha cancellato la regolarizzazione di 20.000 docenti precari già abilitati all'insegnamento? Per non parlare poi delle vergognose parole pronunciate dal ministro Brunetta proprio sui precari, definiti «la peggiore Italia». Che dire, ancora, del Ministro del lavoro che da tre mesi non risponde a una nostra interrogazione sul licenziamento di 1.800 lavoratori in somministrazione dell'INPS, vale a dire di un ente sottoposto alla sua diretta sorveglianza? E ancora: che dire del fatto che vi sono migliaia di vincitori di concorso che non possono veder realizzati i propri sforzi e meriti, quando, peraltro, vi sono in alcuni enti e amministrazioni fabbisogni reali di nuova occupazione? Gli italiani, questa è la verità, con la quale dovrete finalmente fare i conti, hanno capito che questo Governo è arrivato al suo capolinea. Non siete più maggioranza nel Paese, non avete un'idea di come governarlo e cercate di tirare a campare un giorno dopo l'altro, continuando così a far del male all'Italia. La mediocrità del provvedimento che ci accingiamo a votare spiega da sola perché il Paese vi ha sfiduciati e perché non si può andare avanti così. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, nel confronto dialettico tra maggioranza e opposizione sui risultati conseguiti da questo Governo una questione appare assodata. Anche se condita da argomentazioni a volte capziose, come quelle appena svolte dal collega Passoni, infarcite spesso da «però», «si poteva fare di più», «si poteva fare meglio» (perché non basta mai), l'analisi che fa l'opposizione pare non mettere in discussione il consolidamento della stabilità finanziaria, punto che il Governo ha testardamente (ma meritoriamente) mantenuto fermo nella navigazione del difficile, difficilissimo mare che abbiamo attraversato in questi oltre due anni di crisi. Non era così fino a qualche tempo fa. C'è voluto il Presidente della Repubblica per aiutare il Governo Berlusconi a mantenere in ordine quei conti, precondizione necessaria per poter tentare, provare ad avviare politiche di sviluppo e di sostegno all'economia come quelle contenute in questo decreto. Un altro punto assodato è, che la necessità della nostra economia è quella di crescere e l'obiettivo espresso in termini di superamento della crisi può essere raggiunto a patto che vi sia una crescita stabile e duratura che faccia i conti con i rigurgiti di una crisi che cambia faccia

detto, anche in questo nostro sistema economico così frammentario (nel termine positivo del termine), costituito dalla straordinaria presenza di una piccola presenza di una piccola e piccolissima impresa che riesce ad affrontare meglio il primo impatto della crisi in quanto rete, in quanto sistema molecolare che assorbe l'onda d'urto della crisi (che su altri sistemi economici ha invece impattato più improvvisamente e più duramente), noi comunque, nonostante questo, scontiamo il prezzo di alcuni processi mai affrontati con serenità e sincerità, in ordine soprattutto a a quel mercato del lavoro dove ancora i numeri che oggi la crisi mette così tanto in evidenza sono il frutto di una sua rigidità, di una sua pesantezza e soprattutto di una sua conformità ad un sistema ideologico completamente superato, se non spazzato via dalla storia, e dalla storia economica, dei Paesi, dei sistemi occidentali. A me poi A me poi pare evidente che un aumento del tasso di crescita del PIL, a parità di debito pubblico, porti automaticamente ad una riduzione del rapporto tra le due grandezze fondamentali, e anche su questo maggioranza ed opposizione paiono convenire. Cosa ci divide, quindi? Ci divide il "come" il nostro Paese dovrebbe crescere: ricette basate su postulati completamente diversi. Per grandi linee: una che incide sul lato della domanda, volta soprattutto ad incrementare le entrate; l'altra volta a contenere le spese e ad agire sul lato dell'offerta piuttosto che incrementare il gettito, al limite abbassando contemporaneamente entrate e spese, nel tentativo di trovare quel punto di equilibrio che il nostro Governo sta garantendo al Paese. Noi infatti siamo convinti sostenitori del no a nuove tasse e del sì a misure che stimolano l'economia e mantengono il vincolo di bilancio; siamo convinti sostenitori, cioè, di misure che possano innescare quella spirale virtuosa che consente di ridurre il debito e aumentare le risorse a disposizione per la crescita, siano esse di natura pubblica, siano esse di natura privata, come le riduzioni delle imposte o le liberalizzazioni, quelle che facciamo tanto fatica in questo Paese (siano Governi di centrosinistra o di centrodestra) a governare, coperte coperte però, per quanto ci riguarda, non con il ricorso al deficit, ma ad esempio con l'eliminazione di evasioni ed esoneri, o privilegi, oggi ingiustificati. Questo mi sembra l'impianto logico sul quale poggiano i provvedimenti che il Governo, sorretto dalla sua maggioranza, sta elaborando per il semestre europeo, per mantenere quegli impegni così fortemente assunti per la nuova *governance* economica comunitaria. Questo mi sembra il Governo intenda sottolineare quando, nel Piano nazionale delle riforme, mai ricordato abbastanza e recentemente esaminato, considera conclusa l'epoca della politica economica fatta esclusivamente con la spesa pubblica e apre a quella a quella delle misure a basso o nullo impatto sui conti pubblici, ma con effetti significativi sul PIL e sull'economia; in altre parole le riforme necessarie a questo Paese per liberare le proprie energie, per rallentare il corso della crisi, per allentare il morso talvolta troppo stretto di egoismi nuovi o vecchi, di troppi privilegi, di troppe burocrazie. Questo è l'assunto del decreto-legge che andiamo ad esaminare e che andremo a concludere domani con il voto, consapevoli del fatto che questo decreto per lo sviluppo, per quanto qualcuno voglia fare della facile ironia, è un tassello importante per la ripresa dello sviluppo del nostro Paese, che rientra nell'ambito delle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo in tema di risanamento di bilancio e di riforme per Europa 2020. È un provvedimento che è passato un po' in sordina, molto ben lavorato dall'altro ramo del Parlamento, ma completamente coperto dal punto di vista mediatico dalla cosiddetta manovra, il decreto finanziariamente, e quindi mediaticamente, più rilevante varato giovedì scorso.

contiene una folta serie di disposizioni, originariamente proposte dal Governo e integrate, nel corso dell'esame alla Camera, con l'approvazione di emendamenti provenienti sia dalla maggioranza che dall'opposizione, secondo la sana regola di convivenza civile e di grande capacità politica che è quella dell'ascolto e della condivisione. Si tratta di norme che, senza impattare sui conti pubblici, sono volte a stimolare l'occupazione ad aumentare il livello di competitività del nostro Paese. Come inquadrare, se non così, le grandi misure di semplificazione, come quelle in tema di appalti, di cui all'articolo 4, volte a ridurre tempi di realizzazione delle opere pubbliche (uno dei più grandi deficit del nostro Paese) e a semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti, garantendo al tempo stesso un più efficace sistema di controllo e di riduzione del contenzioso? Contenzioso che oramai è il convitato di pietra in ogni bilancio di imprese private che fanno i conti con l'amministrazione pubblica. Come inquadrare, se non così, le misure di liberalizzazione e di semplificazioni e le molte disposizioni in materia di costruzioni private all'interno dell'articolo 5? Una serie di deregolamentazioni in materia di ambiente, appalti, tutela della riservatezza e prevenzione antincendi, a vantaggio di imprese che dovrebbero beneficiare di un alleggerimento nei costi per poco meno di un punto di PIL, secondo una quantificazione recentemente svolta. Altri 7 miliardi annui si affiancano a questi dalla norma taglia-oneri, contenuta in una disposizione ormai per noi lontana, quella del 2008.

più vicino al contribuente-cittadino le misure che questo Governo ha inteso intraprendere in tema di lotta all'evasione fiscale. il Governo perché siamo riusciti, tra il lavoro della Camera e quello del Senato, a riportare al centro del nostro impegno quotidiano, come Governo e come maggioranza, il cittadino che lavora, che paga le tasse e che deve poter continuare ad avere fiducia nel nostro sistema Stato. Signora Presidente, nel mio breve intervento cercherò di richiamare, rispetto al provvedimento in esame recante misure per il Semestre europeo e prime disposizioni urgenti per l'economia,

di appello all'opposizione perché collabori, presenti proposte, dia suggerimenti, si apra al dialogo, se la risposta è sempre questa: no, e ricorso alla fiducia. Credo che ormai sia una menzogna offensiva. Tornando ai rilievi anzitutto al tipo di decreto-legge: 14 articoli delle più disparate materie uniti da un unico elemento di tipo finalistico, cioè l'obiettivo. Ma questo stesso leggero legame non vale per tutte le norme. Ad esempio, non vale per l'articolo 9, che, al comma 3, istituisce una fondazione di diritto privato, a cui parteciperebbero il Ministero dell'economia e il Ministero dell'istruzione. Si trasforma così il fondo per il merito, istituito con la riforma dell'università, che peraltro utilizzava i fondi del diritto allo studio sottraendoli alle università e alle Regioni, per costituire questa fondazione - a mio avviso

sette articoli per infilare qualcosa in questo decreto per lo sviluppo che desse l'illusione di semplificare le procedure per i cittadini e le aziende, non avendo altro di più sostanzioso da immaginare per sorreggere l'economia del nostro Paese.

Lo stesso potrebbe dirsi per la questione della revisione degli appalti, in particolare per la norma che alza il limite per le procedure di pubblica evidenza.

ribasso, che da un lato abbasserà la qualità delle prestazioni che verranno offerte alla pubblica amministrazione e dall'altro permetterà le infiltrazioni, che si vorrebbero impedire con le *black list* inserite in un altro articolo di questo Veniamo poi alle questioni europee. Trattandosi di decreto che nasce dal semestre europeo,

il credito d'imposta per università e ricerca. Come formulata, essa infatti allunga i tempi, perché richiede l'autorizzazione europea per non essere in violazione delle norme sugli aiuti di Stato; inoltre, lavorando sul differenziale,

Molte delle colleghe sono andate ad ascoltare il loro punto di vista, perché abbiamo subito lo scippo dei risparmi realizzati con l'innalzamento dell'età pensionabile per le donne del pubblico impiego. scippo, perché questi soldi, che dovevano essere destinati alle politiche di conciliazione, e quindi a favorire l'occupazione femminile, sono finiti nel calderone del Tesoro. sappiamo che, con la prossima manovra, questa scelta verrà confermata. Intanto, questo è un tradimento dei patti fatti con i cittadini, perché se si dice alle donne italiane

Signora Presidente, colleghi senatori, signor rappresentante del Governo, il decreto-legge oggetto della nostra discussione, efficacemente definito decreto sviluppo, rappresenta un passaggio cruciale, non solo per l'azione di governo, ma per il futuro dell'intero Paese. Le scelte di politica economica che sono state compiute finora hanno mirato a rafforzare la sostenibilità finanziaria del sistema Italia, attraverso un incisivo abbattimento del deficit, nel quadro delle direttive e delle procedure concordate in sede europea. Infatti, insieme alla Germania, in questi anni l'Italia ha ottenuto le migliori *performance* europee per quanto riguarda il rapporto deficit-PIL, grazie ad un programma di rigore e di tagli alla spesa cominciato già dal 2008, con il decreto n. 112, proseguito con il decreto n. 78 del 2010, e che si concluderà con la manovra che a giorni sarà all'esame di questa Camera. Come ben noto, l'obiettivo è l'azzeramento del deficit nel 2014 e il cronoprogramma attuato e da attuare, concordato in sede UE, è riportato in tutti i documenti di programmazione prodotti in questi anni dal Governo e dal Parlamento italiano, l'ultimo dei quali è il recente Documento di economia e finanza, redatto nel pieno rispetto delle regole del semestre europeo. Questo dimostra quanto siano pretestuose le le polemiche di queste ore sulle annualità dei tagli, nella manovra che andremo a esaminare dalla prossima settimana. Nessun Paese in Europa può vantarsi di avere ottenuto risultati migliori dell'Italia; questo ha contribuito a rafforzare la nostra credibilità nell'area euro e a tenerci lontano dai noti e drammatici problemi di altri Paesi europei, nonostante l'Italia avesse condizioni di partenza ben più gravi, soprattutto sul fronte del debito pubblico. È evidente che tale politica di rigore abbia avuto, e abbia tutt'ora, effetti immediati depressivi sulla crescita economica e sullo sviluppo; a voler semplificare, se avessimo scelto di mollare un paio di punti sul deficit, avremmo senza dubbio guadagnato almeno un punto sulla crescita del PIL, ma probabilmente ci troveremmo in ben altri guai. avrebbe visto il nostro Paese essere ancora al di sotto, nel rapporto deficit*-*PIL, rispetto ad importanti Paesi, come la Gran Bretagna e la Francia. È chiaro quindi che è fondamentale mettere in campo politiche che incoraggino lo sviluppo e l'economia, senza d'altro canto cedere alcunché rispetto al rigore della tenuta dei conti pubblici, ma facendo solo in modo di mitigare gli effetti depressivi di tale rigore. Il provvedimento in esame risponde a tale esigenza, in linea anche con quanto indicato nei documenti comunitari a cominciare dal recente Patto Il perseguimento di un risanamento credibile e sostenibile e l'adozione di misure strutturali volte a potenziare la crescita sono priorità fondamentali per tutti, cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Eliminare gli ostacoli normativi e amministrativi, riducendo la pressione regolamentare che condiziona il funzionamento dei mercati, sancire regole più efficaci ed adeguate ad un mondo globalizzato, migliorare il contesto imprenditoriale e i servizi, rafforzare le politiche della ricerca e dell'innovazione, rendendo concrete le misure contenute nel Programma nazionale di riforma e nel Programma di stabilità presentati al Consiglio europeo il 6 maggio scorso, rappresentano obiettivi urgenti ed ineludibili, che trovano conferma anche nel provvedimento in esame. È dunque questo lo spirito che anima il decreto sviluppo, un provvedimento con cui si intende realizzare una serie di misure finalizzate alla crescita e al rilancio dell'economia, in primo luogo attraverso l'istituzione di crediti di imposta a favore delle imprese che investono in misura incrementale rispetto agli investimenti in ricerca nell'ultimo triennio. Al riguardo, non vedo il motivo per cui qualche rappresentante dell'opposizione continua ad insistere sulla presunta penalizzazione delle imprese che hanno investito in ricerca negli anni passati: non è così. Infatti, per quegli investimenti continuerà ad esservi la deduzione dall'imponibile e per gli investimenti incrementali vi

in quella parte del Paese in cui il capitale umano è più a rischio e lo stimolo al mercato del lavoro deve concorrere alla creazione di irrinunciabili condizioni di legalità, necessarie per ridurre il sommerso e quelle disparità territoriali ostative alla realizzazione di pari opportunità per tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui vivono.

a valere sui fondi strutturali, in particolare sul FESR, misura a cui i Presidenti delle Regioni stesse potranno accedere discrezionalmente. Tali disposizioni sono in linea con quanto previsto nel Patto per l'euro, con il quale l'Italia si è impegnata, tra l'altro, a ridurre il differenziale economico tra Nord e Sud,

e il presidente Azzollini - sulla natura solo regolamentare del decreto che andrà a definire i tetti per l'utilizzo dei fondi strutturali europei per questa misura. Ritengo non vi sia alcunché di scandaloso nel fatto che il decreto non sia regolamentare, perché si tratta di stabilire una quota.

La seconda parte del decreto punta ad introdurre norme di semplificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione da una parte, e cittadino ed imprese dall'altra, e alla liberalizzazione delle attività economiche. È l'inizio di uno sforzo importante che Governo e maggioranza dovranno produrre in questa coda di legislatura. Si parte dal rilancio dell'offerta turistica, potenziale di crescita senza eguali per il nostro Paese, introducendo la possibilità di istituire, nei territori costieri, distretti turistici a burocrazia zero, per assicurare alle imprese che vi operano opportunità di investimento, agevolazioni fiscali, finanziarie e amministrative, a beneficio di servizi più efficienti che siano volano di un circuito produttivo virtuoso. In tempi di rigore dunque, lo stimolo alla crescita è l'obiettivo che questo Governo intende continuare a perseguire, ponendosi al fianco delle imprese nella loro faticosa battaglia quotidiana. anche il disegno di modifica al codice dei contratti pubblici, che si prefigge di accelerare le procedure di affidamento degli appalti - soprattutto se si tratta di opere di interesse strategico - e di consentire, da un lato, una rapida cantierizzazione degli interventi infrastrutturali e, dall'altro, una riduzione dell'enorme mole di contenzioso esistente in materia. La proposta di ampliare la discrezionalità delle amministrazioni pubbliche e delle stazioni appaltanti, aumentando la soglia entro la quale è consentito affidare lavori con procedura negoziata e senza bando, non va tuttavia intesa quale rischio a discapito della trasparenza delle procedure di affidamento dei contratti. La concorrenzialità della procedura, con l'aumento del numero minimo dei soggetti che devono essere obbligatoriamente invitati, la verifica dell'esistenza di un adeguato sistema di qualità e dei cosiddetti requisiti di moralità che le imprese partecipanti devono possedere, oltre ad una serie di modifiche e di semplificazioni sulle cause di esclusione dalle gare, contribuiscono a contenere la discrezionalità delle stazioni appaltanti e a garantire l'operatività di un sistema di controllo che renda concreta l'applicazione dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, pari trattamento, trasparenza e proporzionalità. Liberalizzazioni e semplificazioni sono previste anche per quanto concerne l'edilizia privata, con nuove norme che spaziano dall'introduzione del silenzio assenso per il rilascio del permesso di costruire - ad esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali - alla tipizzazione di un nuovo schema contrattuale al fine di conferire certezza alla diffusa prassi della cessione di cubatura. E ancora, l'istituzione di una fondazione per il merito, per concedere prestiti agli studenti più meritevoli, un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, un fondo rotativo per il sostegno a imprese e ricerca, lo snellimento degli adempimenti degli adempimenti di natura fiscale nelle operazioni di rinegoziabilità e portabilità dei mutui, fino ad una modifica nell'ambito di applicazione del codice della *privacy*, con l'obiettivo di eliminare oneri inutili sul piano pratico e ingiustificati ai fini della tutela dei dati, costituiscono tutte misure idonee a configurare un unico disegno: ridurre i costi e i carichi derivanti da vischiose pastoie burocratiche, a beneficio di uno Stato apparato più moderno, che non condanni la comunità civile a un'inesorabile stagnazione ma che sia, al contrario, garanzia di una maggiore coesione sociale e una più alta qualità di vita. Sud)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, parola nel contesto degli interventi dei colleghi dell'intera opposizione e, più in particolare, del mio Gruppo, quindi non condurrò un esame generale di questo provvedimento, perché sarebbe inutilmente troppo complicato e troppo lungo.

Ritengo che questo provvedimento parli ben poco di sviluppo e pratichi molto, ma molto, di degrado. Gli articoli 4 e 5 lo dimostrano in maniera abbastanza significativa. Siamo di fronte ad una logica che impone il primato della deroga. Se si legge riga per riga nei particolari questo provvedimento, si scopre che, di volta in volta, man mano che va avanti, sui singoli punti di interesse del provvedimento si stabiliscono deroghe alle leggi precedenti, leggi che qualche volta erano più vincolanti, qualche volta magari poco chiare, ma comunque tentavano di determinare una sorta di effetto di controllo soprattutto sui beni di interesse pubblico. Nel decreto, invece si registra questo primato della deroga, che si esercita puntigliosamente nello scardinare la possibilità di controllo sulla gestione dei beni di interesse pubblico.

alle conseguenze sul panorama territoriale italiano. Voglio dire ai colleghi, per cominciare, una cosa molto semplice: basta che ognuno di loro vada a vedersi le carte geografiche, le foto aeree dell'Italia degli anni '50, appena uscita dalla guerra, e le foto aeree dell'Italia all'inizio di questo secolo, per verificare da solo, anche senza essere né urbanista né geografo, una cosa di elementare semplicità: semplicità: i centri storici di una volta sono diventati entità estremamente ridotte, conchiuse ed accerchiate da una panorama di estensione urbanistica di proporzioni stupefacenti.

La campagna è stata vigorosamente urbanizzata nelle maniere più insensate, moltiplicando zone che apparentemente avevano all'inizio qualifica di strumenti dello sviluppo economico e che si sono rilevate sostanzialmente occupazione occupazione di suolo, insensata, dissipata, senza risultati economici, spesso con il solo degrado del quadro fisico italiano. Esistono pezzi interi di Italia, dove l'insediamento storico rifuggiva dalla presenza lungo la costa per tradizioni antiche, popoli pastorali, agricoli, che non avevano nessun interesse al mare, e che oggi presentano, agli occhi più o meno stupefatti di chi vada a vedere la situazione, città lineari, costiere senza soluzione di continuità che legano comune a comune e moltiplicano, certe volte per due o per tre, i paesi che stavano nell'interno e che oggi sono diventati paesi costieri. Tutto ciò è stato realizzato, tra l'altro, con una qualità edilizia in generale abbastanza scadente, perché le esigenze della ricostruzione *post*-bellica hanno costretto i soggetti - cosa comprensibile - a tirare via a costruire, ricostruire, spesso con

decreto prenda in esame questa situazione e cerchi di porre rimedi; si scopre invece che i rimedi sono peggio del male, perché il primato della deroga determina sostanzialmente un «liberi tutti»: si può fare qualsiasi cosa. Sono già stati citati esempi che rimarranno di scuola, tipo l'allungamento di venti anni del limite dell'età ragguardevole per meritare il titolo di edificio o struttura da salvaguardare, che passa quindi dai 50 ai 70 anni. Può sembrare uno scherzetto; in fondo, che saranno mai vent'anni! Se uno va a vedere la

spostare il confine della salvaguardia dai 50 ai 70 anni determina degli effetti che potrebbero essere scandalosi. Edifici che oggi vengono visitati dagli studenti, e magari persino dai turisti, in qualche caso, potrebbero risultare come indifendibili, perché tanto ormai stanno all'interno del confine dei 70 anni e quindi non sono più proteggibili come avrebbero potuto essere secondo le normative precedenti. L'uso disinvolto, ai limiti della nequizia, del federalismo demaniale produce delle mostruosità. Per esempio, la

Secondo il codice Urbani, articolo 146, comma 5, il parere del soprintendente sulle autorizzazioni paesaggistiche era vincolante in prima applicazione ma diventa obbligatorio dopo che i vincoli paesistici sono stati incorporati dagli strumenti urbanistici di piano. In questa maniera non risulta più vincolante e funziona il criterio temibilissimo del silenzio assenso, un'espressione che i parlamentari affezionati ai beni comuni del territorio e del paesaggio dovrebbero sentire pronunciare solo con i capelli ritti. Tale principio consiste nel fatto che, se l'autorità pubblica non risponde entro un limite determinato, il silenzio vale come assenso.

si può fare qualsiasi cosa. Direi che sul tema si dovrebbe fare una riflessione di natura costituzionale, perché

purché non sia in contrasto con l'utilità sociale. So bene che la maggioranza punta a erodere questa piccola espressione «in contrasto con l'utilità sociale», che dà una noia terribile. Il centrodestra ne ha fatto una bandiera di questa lotta: togliere dall'articolo 41 della Costituzione il limite del contrasto con l'utilità sociale. In questo caso, però, mettiamo in mano al roditore privato, o meglio alla platea non esigua dei roditori privati, la possibilità di incidere su un

cui veramente si tocca con mano il capovolgimento totale del paradigma. Quello che passa come riqualificazione urbana e rinnovamento della città prevede una volumetria aggiuntiva premiale per chi interviene sulla modifica della struttura edilizia preesistente; prevede la delocalizzazione, la possibilità di prendere un volume che sta in un punto e spostarlo da un'altra parte; prevede inoltre il cambio di destinazione d'uso, le modifiche della sagoma; prevede che gli immobili abusivi, inclusi in una sorta di titolo abilitativo in sanatoria, siano tranquillamente salvati;

prevede - fissazione ontologica di questa maggioranza parlamentare - un'ulteriore esaltazione dei poteri dell'Esecutivo. Infatti, sulla possibilità di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (ripeto il termine, che però è presente nella legge: si costruisce in deroga agli strumenti urbanistici),

fondamentali che dovrebbero insistere sulla salvaguardia del paesaggio e del territorio passano in mano alla Giunta. Mi rendo conto che sto parlando di cose che alla maggioranza interessano poco, ma noi dentro questo provvedimento, apparentemente così allargato a tutto il ventaglio delle iniziative per lo sviluppo, stiamo ponendo esclusivamente la possibilità dello sviluppo edilizio. Ho detto all'inizio che la Repubblica italiana ha già conosciuto uno sviluppo edilizio insensato, ipertrofico e tra l'altro privo persino in molti casi di redditività economica:

sono solo in attesa di compratori e affittuari che non arrivano mai. A cosa servono? Ve lo dico io, ma gli specialisti lo sanno: servono ad accenderci ipoteche. Oggi in Italia possedere un capannone è un mezzo per avere soldi dalle banche: il capannone non serve a niente, non ci lavora dentro nessuno, nessuno porta materiale

purtroppo con il tutto. Stiamo consumando il bene finito del territorio e del paesaggio in modo insensato, dissipativo, senza rispetto per la logica costruttiva del passato e per le attese delle generazioni che verranno. Stiamo facendo un errore di natura veramente epocale (questo sì davvero epocale) e purtroppo noi, che siamo minoranza, non riusciamo a impedirlo, però nutriamo la ragionevole speranza che questa epoca così avvilente della Repubblica italiana sia lì lì per finire*.

non sono andate probabilmente nel segno desiderato da parte della maggioranza. Alcune questioni sono state risolte, ma io mi volevo soffermare su altre che presentano ancora delle grosse criticità,

particolare. Il decreto interviene, per esempio, sulle principali criticità relative alla normativa sulla riscossione, ma non appare risolutivo e rispondente alle aspettative di riforma, alimentate peraltro dagli impegni recentemente assunti in sede parlamentare e dalle dichiarazioni pubbliche rese da alcuni dei maggiori esponenti dell'Esecutivo. Per questo risulta importante, e a mio giudizio risolutivo, un ordine del giorno che è stato presentato alla Camera dei deputati dal Gruppo di Futuro e Libertà, e che il Governo ha accolto,

al suo impegno, di effettuare una ricognizione complessiva della normativa in materia per introdurre norme che permettano: il superamento del principio del *solve et repete*, contrario ai principi costituzionali di garanzia e di presunzione di innocenza (a partire dall'abolizione della norma sull'immediata esecutività degli avvisi di accertamento); l'allungamento dei piani di rateizzazione e abolizione degli interessi di mora per i contribuenti a più basso reddito; la revisione degli studi di settore per le imprese; l'individuazione di paletti per Equitalia e gli altri agenti della riscossione in materia di interessi di mora, di sanzioni e di aggio della riscossione applicabili. applicabili. Tutto questo per rivedere in termini più equilibrati il rapporto tra cittadino contribuente e Stato e per dedicare una maggiore attenzione ai cittadini a più basso reddito;

è ancora tutto sul piatto, è quello relativo ai crediti verso la pubblica amministrazione. I crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione ammontano a circa 60 miliardi di euro l'anno; l'abbiamo detto in questi mesi e in questi anni, non so quante volte l'abbiamo ripetuto e abbiamo sollecitato l'attenzione I tempi della solvibilità dello Stato verso i suoi fornitori nel 2010 si sono allungati fino a 186 giorni lavorativi; si tratta di cifre distanti dalla media degli altri Paesi dell'Unione europea. Questi ritardi rappresentano un problema enorme per le nostre imprese e sono all'origine di un fallimento su quattro e della perdita di 450.000 posti di lavoro all'anno. Questi ritardi compromettono il corretto funzionamento del mercato interno e costringono le piccole imprese a ricorrere a finanziamenti esterni che riducono le loro possibilità di investimento e ne minano quindi la competitività. In un periodo di regressione economica le conseguenze possono essere ancora più gravi, a causa anche delle difficoltà di accesso al finanziamento, di cui parlerò dopo in relazione ad un altro articolo che è stato inserito nel decreto sviluppo (l'articolo 8-*bis*). Dobbiamo ricordare che l'Italia resta sotto esame da parte delle agenzie di *rating*, dopo il monito di Moody's e di Standard and Poor's, che hanno peggiorato le prospettive sul merito

proprio questo tema. Tale emendamento prevedeva da una parte l'istituzione di una società presso la Cassa depositi e prestiti dedicata allo smobilizzo dei crediti che le piccole e medie imprese vantano nei confronti delle pubbliche amministrazioni

questo. Se ci sono due Camere, facciamole funzionare e facciamo in modo che quello che si può migliorare venga migliorato. Sarebbe stato comunque possibile osservare la scadenza del decreto, pur

di smobilizzare il credito presso il sistema bancario. Si tratta quindi di un tema centrale, di cui parliamo da anni e che è ricorso negli interventi di chi mi ha preceduto, ma che è

Tra le conseguenze della modifica approvata alla Camera dei deputati vi è l'eliminazione di una parte importante delle informazioni creditizie oggi disponibili, a dispetto di quanto previsto dalla regolamentazione di settore, cioè dal codice di deontologia e di buona condotta per i

l'ipotesi di modifica di questa normativa costringerà banche ed intermediari finanziari ad attuare politiche di erogazione del credito fortemente prudenti. Pertanto, si avranno ulteriori ripercussioni per le piccole e le medie imprese che non potranno neanche smobilizzare i crediti verso le pubbliche amministrazioni; infatti, il sistema bancario chiederà garanzie aggiuntive perché non avrà più la cosiddetta storia creditizia e quindi non sarà più in grado di distinguere i soggetti affidabili da quelli che non lo sono. Questo paradossale ma inevitabile effetto restrittivo penalizzerà soprattutto i consumatori che sono virtuosi, cioè i buoni pagatori, e nel contempo favorirà comportamenti sleali da parte dei richiedenti credito non intenzionati ad onorare gli impegni assunti. Allora, attraverso altri strumenti, come le moratorie sul credito, si possono raggiungere i desiderati obiettivi di facilitare l'uscita dalla crisi per i consumatori e le imprese che hanno difficoltà a rimborsare i finanziamenti. È stato accolto dal relatore e dal ordine del giorno a mia firma con cui si chiede di rivalutare il problema individuando soluzioni realmente efficaci per il sostegno delle persone fisiche e giuridiche che scontano la reale congiuntura economica e di adottare iniziative normative che riconsiderino le modifiche introdotte dall'articolo

di un Governo che governi, con la priorità del risanamento dei conti pubblici e della crescita, altrimenti non si crea ricchezza ed occupazione.

e sul quale credo che tutti noi, sempre di più, insisteremo fintanto che non otterremo la reale, giusta attenzione da parte del Governo in questa occasione e nel dibattito che si aprirà la prossima settimana sulla manovra finanziaria.

e di danno, perché sono norme che, da una parte, recheranno un danno grave alla tutela del nostro patrimonio ambientale e paesaggistico e dei nostri beni culturali e, dall'altra, non faranno risparmiare un euro alle casse dello Stato e non avranno alcuna utilità dal punto di vista del rilancio dello sviluppo. Parto dalla prima di queste norme, contenuta nell'articolo 4, che riguarda l'azzeramento del carattere vincolante delle autorizzazioni paesaggistiche in capo alle soprintendenze per quanto riguarda le opere pubbliche, quelle strategiche ma anche quelle di più modesta dimensione.

da chi governi, sia di destra o di sinistra, soprattutto in un Paese come il nostro dove il paesaggio e i beni culturali sono un elemento fondante sia dell'identità nazionale, che di una parte non piccola del PIL. Secondo uno studio presentato dalla Fondazione Symbola pochi giorni fa, l'economia direttamente legata a questi settori vale oltre il 5 per cento del nostro prodotto interno lordo. In questo cosiddetto decreto sviluppo l'articolo 5 riguarda la liberalizzazione delle costruzioni private. Si tratta dell'ennesimo piano casa che introduce il silenzio assenso per i permessi di costruire e allarga ulteriormente gli ambiti di applicazione SCIA, la la segnalazione certificata di inizio attività, in forza della quale si possono aprire cantieri per piccole e grandi ristrutturazioni senza neppure aspettare che scadano i termini del silenzio assenso. Come gli altri piani casa, anche questo è destinato a non produrre alcun effetto anticiclico, ma evidente ragione che, se in Italia l'edilizia ha problemi, non è per un eccesso di regole, ma per la crisi. I dati dimostrano che l'Italia negli ultimi dieci anni è stato uno dei Paesi europei dove si è costruito di più.

Se l'edilizia oggi in Italia è in difficoltà - ripeto - è a causa della crisi, e anche di un modello di sviluppo territoriale che da una parte massimizza il consumo di suolo e dall'altra non affronta il vero nodo del disagio abitativo che è la mancanza di un accessibile e rilevante mercato degli affitti. Questa norma, come gli altri piani casa, non produrrà dunque alcun rilancio dell'edilizia: semmai incoraggerà ancora di più quel fai da te edilizio e urbanistico che in Italia, Paese leader in Europa per il mattone abusivo, ha già provocato tanti scempi. La nostra idea per rilanciare l'edilizia è alternativa alla vostra. Per esempio, vi è la proposta con cui abbiamo chiesto e chiediamo da tempo (nella discussione di questo provvedimento, con la sostituzione dell'articolo 5) di stabilizzare il credito d'imposta del 55 per cento per le ristrutturazioni energetiche delle abitazioni, che scade il prossimo 31 dicembre. Una misura introdotta a suo tempo dal Governo Prodi che voi avete tentato di cancellare e avete, comunque, depotenziato, portando da 5 a 10 anni il periodo in cui spalmare le detrazioni fiscali. Un incentivo, questo sì, davvero anticiclico, che ha incontrato nei quattro anni in in cui è stato in vigore uno straordinario successo: un milione di cantieri aperti, 11 miliardi di fatturato, un risparmio energetico pari all'energia prodotta in un anno da una grande centrale termoelettrica. Con i *referendum* di poche settimane fa la maggioranza degli italiani (non solo di sinistra, perché è stato calcolato che a quei *referendum* hanno partecipato almeno 8-9 milioni di elettori di centrodestra, che erano, sono e magari rimarranno io spero di no - elettori di centrodestra) ha chiesto alla politica di occuparsi di più e meglio dei beni comuni e, attraverso i beni comuni, del bene comune. Se il decreto che voi chiamate sviluppo è la risposta a questa domanda, credo che esso, anche nelle parti che riguardano la tutela del paesaggio e il governo del territorio, sia la prova ormai lampante che questa maggioranza e questo Governo hanno perduto ogni capacità di preoccuparsi e di occuparsi dei veri interessi e dei veri bisogni del nostro Paese.

forse questo dibattito potrebbe apparirci inutile, stretto com'è tra l'ennesimo voto di fiducia e la manovra imponente che verrà in discussione dalla prossima settimana. Penso invece che questo dibattito serva a qualcosa: secondo me a dimostrare ancora una volta l'immobilismo del Governo. Il tempo dell'azione, che sarebbe così prezioso in un momento di crisi rilevante come quella che attraversiamo, viene disperso da un Governo che non sa o non può assumere delle decisioni riformatrici. È perciò un altro semestre perso: era di dicembre la promessa fatta in quest'Aula dal Presidente del Consiglio di un nuovo inizio e l'annuncio in gennaio di un decreto che sarebbe stata la frustata più grande mai vista dall'economia italiana. La frustata si è ridotta a questo decreto debole e timido. Penso che sia una costante dell'azione del Governo in questa legislatura. Se qualcuno avesse la curiosità (i colleghi o anche i cittadini che ci stanno ascoltando) di rileggere il dibattito sulla prima manovra economica di questa legislatura, nel luglio 2008, potrebbe vedere un'opposizione che già allora denunciava con chiarezza il carattere strutturale della crisi, la sua profondità e la necessità di adottare subito misure per lo sviluppo e la difesa dei redditi, ma vedrebbe anche la sordità totale della maggioranza. Signor Sottosegretario, non sono tra quelli che criticano il Governo perché il grosso della manovra correttiva è collocata nel 2013 e nel 2014. Non lo faccio per due motivi: perché nel 2011 e nel 2012 agiscono e agiranno i pesanti tagli previsti dal precedente decreto del 2010, cosa che molti sembrano dimenticare, ma di cui sono ben coscienti ad esempio i nostri sindaci; poi perché in un clima economicamente depresso non bisogna aggravare le tendenze recessive. Tuttavia questa scelta avrebbe dovuto portarne con sé un'altra: utilizzare tutto questo tempo, e avreste dovuto farlo fin dai primi giorni della legislatura, per una decisa azione riformatrice; utilizzare il tempo per incardinare quelle riforme che possono costare nell'immediato, ma che producono maggiore crescita nei tempi medi o che sono a costo zero, ma richiedono un po' di tempo per produrre effetti. Nulla di tutto questo. Mi limito a sottolineare tre aspetti. In primo luogo, il credito d'imposta per la ricerca: ottima la priorità, ma discutibile la realizzazione. Il credito d'imposta in particolare per il sostegno alla collaborazione tra università e impresa era stato introdotto dal Governo Prodi nel 2006: lo avete eliminato; l'anno scorso avete stanziato 100 milioni di euro restati senza normativa applicativa: ora finalmente correggete l'errore, ma commettendone un altro. Così com'è scritta la norma, si otterrebbe questo paradossale risultato: l'impresa che in anni di difficile crisi ha stretto i denti e ha continuato a investire in ricerca non avrebbe alcun vantaggio. Ad esempio, ha investito il 5 per cento del fatturato nel triennio 2008-2010 e intende continuare a farlo nel prossimo biennio? Lo Stato non le ha dato niente allora e non le darà niente nel futuro, perché incentiva solo l'incremento dell'investimento. Un'altra impresa ha effettuato zero investimenti nel periodo di crisi e inizia oggi ad investire: tra 90 per cento del credito d'imposta e vigenza della deducibilità, potrebbe addirittura incassare più di quello che ha speso. Non ci sembra il modo migliore di incoraggiare i comportamenti virtuosi delle imprese. Nel settore degli appalti si introducono anche norme positive, tendenti a combattere l'eccesso di ribasso, ad introdurre migliori forme di pubblicità, e così via, ma poi tutto casca sulla scelta di fondo, che è sbagliata: invece di affrontare le ragioni strutturali dei ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche (eccessi di litigiosità, utilizzo ingiustificato di varianti, eccessiva durata delle esecuzioni, insufficiente qualificazione dei soggetti) si sottrae alla concorrenza e a procedure competitive pressoché l'intero comparto degli appalti con la pubblica amministrazione, come ha ricordato ha ricordato il senatore Agostini. Un comparto che vale l'8 per cento del PIL. In questo modo si favoriscono fenomeni corruttivi e amicali, che indeboliranno la capacità concorrenziale dell'industria italiana. Pertanto, l'esito inevitabile sarà che i grandi appalti saranno vinti dalla concorrenza estera e il nostro settore delle costruzioni sarà ulteriormente indebolito. Ma davvero pensiamo che il futuro di un settore così importante dell'economia possa essere affidato ad un contesto senza concorrenza e a imprese che si specializzano nella conoscenza del mercato locale piuttosto che in una capacità competitiva a largo raggio? Potrei perfino comprendere una norma a tempo, con la finalità di dare per quest'anno una straordinaria accelerazione alla committenza locale: ma quale committenza, se il Patto di stabilità stupido impedisce agli enti locali di fare investimenti? E del resto, sul piano della concorrenza, delle liberalizzazioni e delle semplificazioni (ecco le famose riforme a costo zero) i contenuti del decreto sono del tutto carenti. Basta riandare alle parole del professore Catricalà, nell'ultima sua relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato: un grido d'allarme sul completo abbandono di una seria politica di sviluppo di un mercato ben regolato, a cominciare dalla mancanza della legge annuale per la concorrenza, prevista e mai presentata. Infine, è certamente meritoria l'intenzione del Governo di agire sull'eccesso di intermediazione politica e sull'elefantiasi di apparati pubblici e parapubblici dipendenti dal sistema del potere politico centrale o locale. Il problema è che resta un'intenzione,

Ma e soprattutto, mentre si annunciano cose che non ci sono, si fanno le cose che non si dovrebbero fare. Questo decreto darà un bell'impulso alla moltiplicazione di enti pubblici. Infatti, si prevede una Fondazione per il Merito, con la partecipazione di tre Ministeri. Si prevede nientemeno che un nuovo Ente nazionale per il microcredito, con il suo consiglio di amministrazione, la sua dotazione di personale. Togliendo ad Equitalia la riscossione coattiva e riportandola in capo ai Comuni si genererà la costituzione di centinaia di gestioni comunali *in house* o di affidamenti che in passato avevano già mostrato tutti i loro limiti. Ci saranno più enti pubblici, meno riscossioni, più costi di esazione, meno efficienza. E dunque anche per questa via il decreto rende palese il limite sostanziale di questo Governo. Non sono solo i soldi che mancano: questo sarebbe un vincolo per chiunque governasse, anche per noi. Manca invece la visione generale delle condizioni in cui un Paese può crescere: mercati aperti, merito, legalità, buona amministrazione, equità fiscale, formazione del capitale umano e del capitale fisico. Manca l'azione ostinata, ancorché difficile, perché queste restino le bussole dell'azione quotidiana del Governo, perché si trasmetta al Paese un messaggio univoco, un appello alle migliori energie. Manca insomma una visione profondamente riformatrice, quella che il Presidente del Consiglio in verità aveva offerto all'opinione pubblica all'inizio della sua attività politica nel 1994. Ora il grande imbroglio si è pienamente palesato all'opinione pubblica, e anche questo decreto, purtroppo, lo conferma.

una premessa che credo debba essere ricordata da tutti quando affrontiamo simili problematiche. Continuiamo a vivere una crisi finanziaria ed economica che è la più terribile degli ultimi sessant'anni. Qualcuno forse nel 2008, quand'è fallito il più evoluto, moderno e avanzato sistema finanziario del mondo, quello statunitense, s'era illuso che questa crisi avrebbe portato conseguenze per sei mesi, o forse un anno. Così non è stato, e dobbiamo prendere atto che ancora oggi siamo immersi nella più drammatica crisi che mai sia capitata nell'Occidente moderno. In questa situazione, il Governo Berlusconi ha reagito - a mio avviso - per i primi due anni manifestando senso di responsabilità e praticando convintamente una politica di rigore nell'uso delle risorse pubbliche, cioè tenendo a posto i conti pubblici, considerato che abbiamo questa questa zavorra del debito pubblico, che ci appartiene, perché appartiene alla storia di tutti noi. Essendo stato parlamentare anche nella prima Repubblica, ricordo sempre che negli anni '80 nessuno in Parlamento faceva presente che la spesa pubblica eccessiva avrebbe causato di lì a qualche anno le conseguenze che abbiamo visto. Eravamo tutti convinti che la socialità applicata alla gestione dell'economia, soprattutto delle partecipazioni statali, fosse una linea vincente, e lungo questa strada anzi l'appellativo dei migliori e dei più progressisti se lo conquistarono sul campo le amministrazioni di sinistra, che diedero un grande contributo allo sfondamento dei bilanci pubblici di quel tempo. Ciò detto, il Governo ha praticato questa politica

per tutelare i lavoratori fuori del ciclo produttivo messi in cassa integrazione in maniera mai vista nella storia di questo Paese. Quest'anno siamo arrivati al terzo anno della crisi, e il Governo ha capito che ha capito che il rigore fine a se stesso non ci porta da nessuna parte. Se questo Paese non torna a crescere, potremmo sì vantarci di avere i conti a posto, però saremmo il fanalino di coda.

Semplicemente, noi che veniamo da lontano sappiamo che nel nostro Paese la paralisi nelle opere pubbliche ha una data e un nome. La data è il 1993, e se andate a leggere le statistiche (non i bollettini del PdL, ma le statistiche), scoprirete che nel nostro Paese abbiamo realizzato grandiose opere pubbliche

Nel 1993 è però accaduto un fatto clamoroso. La cosiddetta rivoluzione di Tangentopoli ha generato la legge Merloni: un disastro! La legge Merloni è all'origine della paralisi, scientificamente provata,

abbiamo intrapreso il corredo normativo, realizzando tre leggi importanti: la legge obiettivo, il decreto attuativo della legge obiettivo e la legge n. 166 del 2002. E a fine legislatura abbiamo dotato il Paese, primo in Europa, del codice degli appalti, bruciando 57 leggi preesistenti.

in Italia, la maggior parte degli appalti viene assegnata al massimo ribasso. Dopodiché, tutti urlano allo scandalo perché arrivano imprese, (quelle che non pagano i contributi, che non pagano i lavoratori, quelle che oggi nascono e domani muoiono) che vincono gli appalti e poi lasciano incompiuta

utilizza tutti gli spazi di libertà che l'Europa ci consente. Con questo decreto, invece, compiamo questa operazione. Bisogna dunque responsabilizzare le stazioni appaltanti e fare in modo che decidano loro, valutando il prezzo e la qualità del progetto, se è un progetto serio o se espone a rischi non ben identificati. Secondo noi, questo è un tentativo da fare. Sono troppo le stazioni appaltanti in Italia? Certo, sono troppe, e allora il problema è di aggregare le stazioni appaltanti e di convincere il piccolo comune che, se non è in condizione

Noi abbiamo superato tutto questo e abbiamo stabilito che i vizi emendabili si possono emendare. Quindi, abbiamo stabilito una regola in forza della quale riteniamo che gli appalti, dopo la conversione in legge di questo decreto, potranno procedere in maniera molto fluida. In terzo luogo, nel nostro Paese cresce una linea di lavoro che sta prendendo fortemente piede, ed è una linea di lavoro che immagina che soggetti progettino, costruiscano e gestiscano opere pubbliche. Quali? Tutte le opere pubbliche. Tutte le opere pubbliche in grado di generare reddito, dal ponte sullo Stretto di Messina all'autostrada, al termovalorizzatore, alla piscina, al parcheggio, all'ospedale (arriveremo a realizzare anche le carceri) possono - devono secondo noi - essere progettate, costruite e gestite dai privati. E questi ultimi devono capire

I privati devono capire che nascerà una stagione in cui avremo una borsa del mercato delle aziende che gestiscono le opere pubbliche e quindi le aziende più competitive saranno quelle che sapranno gestire le opere pubbliche (un parcheggio, un'autostrada, un termovalorizzazione, una piscina, un porticciolo o quant'altro).

questo provvedimento abbiamo fatto un passo avanti, abbiamo inventato - e speriamo che dopo il plauso delle associazioni di categoria anche i Comuni lo apprezzino - il *project* di terza generazione. Che cosa è il *project* di terza generazione? Oggi un privato per realizzare un parcheggio con la finanza di progetto

secondo una logica di centrodestra, che privilegia, in base a quanto scritto nella nostra Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale, l'iniziativa del privato rispetto alla presenza del pubblico.

rispettasse le leggi e le procedure che deve rispettare una petroliera quando entra in un porto. Abbiamo modificato anche questa normativa, in maniera tale che l'Italia, primo produttore nel mondo di *super-yacht,* che generano ricchezza, anziché assistere impotente a quanto è accaduto l'anno scorso dopo quella vicenda, (tutti i *super-yacht* sono andati a rifugiarsi in Costa Azzurra, in Corsica e in Spagna) li veda ritornare per portare ricchezza all'erario italiano. Queste norme riformano la nautica, come già si fece nel 2002 quando il settore era in crisi e noi, con la legge organica sulla nautica, abbiamo ridato slancio ad un settore che genera ricchezza. Non mi pare che questi interventi siano di second'ordine: essi incideranno sul tessuto economico del nostro Paese, e credo siano il primo serio e costruttivo contributo che il Governo dà ad una politica mirata allo sviluppo e alla crescita, che oggi anche per noi è la regola fondamentale, perché il rigore fine a se stesso non ci porta da nessuna parte.

forse è - io sono per questa terza ipotesi - un progetto da riempire con altre, molte priorità? Vorrei ricordare che un decreto che parla di semestre europeo, disposizioni urgenti per l'economia e di piani di sviluppo a tutto campo, forse è un orizzonte talmente vasto che autorizza anche priorità finora non trattate dai molti interventi fin qui ascoltati. Io ne ho una che non è nuova per quanto mi riguarda, ossia quella della montagna. A costo di apparire monotono, ripeto l'eterno ritornello in ogni occasione che si presta per ricordare che esiste questa priorità, che esiste questa specificità

la prima è la Carta costituzionale italiana, che, all'articolo 44, impone lo sviluppo delle zone di montagna; la seconda è la Carta costituzionale europea,

occorre promuovere uno sviluppo armonioso per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, mirando a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. In questo articolo 174 si esemplifica quali siano considerate in Europa le regioni meno favorite. Si parla di zone rurali, di zone interessate da transizione industriale, di regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, per arrivare alle regioni insulari, transfrontaliere e, finalmente, regioni di montagna. Dico finalmente perché questa specificità finora non era riconosciuta. Dobbiamo al Trattato di Lisbona, quindi al 2009, il fatto che, accanto alle isole, sia stata inserita la montagna come come territorio idoneo ad essere considerato specificità agli effetti dell'utilizzo di incentivi, con deroghe possibili al regime degli aiuti di Stato e delle regole della concorrenza.

al signor Sottosegretario che l'ennesimo appello a tenere in considerazione la specificità della montagna in interventi come questo non è più soltanto una speranza o una pia illusione di coloro che vivono in montagna o che l'hanno a cuore. Vorrei infatti infatti ricordare che più o meno tutti o quasi gli italiani hanno un piede o una radice in montagna, visto che il territorio nazionale è considerato almeno per il 60-65 per cento montano, che ci vive una

questo motivo di attenzione per la montagna ricordando l'articolo 174, che impone attenzione nel settore della coesione regionale per queste zone,

Dico questo perché, purtroppo, anche in questo caso, come in altri, non sono molti i punti di attenzione riservati alla montagna. Si sono andate a cercare specificità Si sono andate a cercare specificità marine, specificità di terreni in degrado, ma per la montagna vi sono un paio di passaggi molto tiepidi. L'articolo 6, comma 2, lettera *b)*, quando parla di obblighi delle pubbliche amministrazioni, tra le definizioni funzionali ricorda che esistono le comunità montane, i loro consorzi e le associazioni; inoltre l'articolo 7, comma 3-*bis*, dove si parla di caratteri di ruralità ai fini fiscali per costruzioni, ricorda che vi sono costruzioni destinate

che fra gli enti di ricerca viene soppresso l'EIM, Ente italiano per la montagna, ex Imont, un istituto di ricerca che aveva

partendo sempre dal presupposto delle Carte costituzionali italiana ed europea, che in questo momento presso la 5a Commissione bilancio è depositato il disegno di legge n. 2566, che abbiamo appena ricevuto dalla Camera dei deputati, il cui titolo è «Disposizioni a favore dei territori di montagna», che ha cominciato in maniera a quanto pare promettente il proprio *iter*.

potrebbe sostituire l'attesa riforma della legge n. 97 del 1994. Ci sono qui al Senato depositati almeno tre o quattro disegni di legge che attendono di essere esaminati, il cui *iter* non è ancora cominciato. Pare non sia il momento favorevole per proporre tutto quello che questi disegni di legge contengono, in termini soprattutto di impegno finanziario, mentre il disegno con sei piccoli poveri milioni di euro, potrebbe cominciare a far capire alla montagna che vi è ancora la volontà ed il desiderio di occuparsi di lei. Questo è un ordine del giorno che sarà proposto all'approvazione dell'Assemblea e che impegna il Governo innanzitutto a ribadire la specificità della montagna, chiede una fiscalità di vantaggio per le zone di montagna, soprattutto per determinate attività economiche in cui, per esempio, i costi del riscaldamento, del gasolio, della elettricità, dell'energia in genere rappresentano un *handicap* nei confronti di altri territori; territori; ma ancora si chiedono iniziative tese a potenziare interventi per la difesa e la conservazione dell'ambiente, l'implementazione di incentivi a favore della multifunzionalità, e soprattutto per le professioni di montagna, per coloro che intendono rimanere a vivere e a lavorare in montagna, garantendo loro magari un reddito dignitoso, competitivo, pari a quello che potrebbero trovare andando a lavorare in città. Ma naturalmente l'obiettivo principale rimane sempre quello di evitare l'abbandono, l'esodo dalle zone di montagna, che significherebbe la perdita totale del sistema montagna,

ha obiettivi di grande respiro e quindi non soltanto di tipo politico, riguarda la difesa di 82 posti di lavoro, di operai stagionali nel Parco nazionale dello Stelvio,

tassarsi, di mettere a disposizione i fondi necessari per compensare la perdita di reddito che queste persone avrebbero con l'approvazione della nuova Si chiede soltanto di onorare gli impegni, e soprattutto di consentire al consorzio del Parco nazionale dello Stelvio di avere l'autorizzazione per applicare questo impegno che, tra l'altro, si risolve a costo zero per il bilancio dello Stato.

pur in una situazione innegabilmente di emergenza come molti colleghi hanno ricordato, accanto a un'attenzione generale per interessi condivisi e collettivi non si possono assolutamente dimenticare incentivi e iniziative a favore di zone forse periferiche, magari meno abitate rispetto alle grandi città, ma che proprio per questo hanno bisogno di segnali più precisi e forse più convinti, che si chiamano solidarietà.

quando abbiamo letto che nel titolo questo provvedimento riportava la dicitura «Prime disposizioni urgenti per l'economia», avevamo sperato che finalmente si volesse aprire un confronto di merito su alcune questioni fondamentali e strutturali che riguardano il futuro dell'Italia. abbiamo scorso il testo aspettandoci di trovarvi qualcosa che, non dico modificasse l'articolo 41 della Costituzione, ma comunque avesse a che fare con quel principio, sempre più invocato, che tutto è possibile salvo quello che non è proibito, applicato almeno alla libertà d'impresa delle medie e piccole imprese, degli artigiani e della ricerca. Purtroppo non c'era niente di tutto ciò. ciò. Noi prendiamo spesso sul serio il Ministro dell'economia, al quale riconosciamo alcuni meriti, almeno nel tentativo di difendere una linea rigorista sui saldi del nostro Paese, e sappiamo che a volte mantiene ciò che dice. Ad esempio, ricordiamo con esattezza che nel corso della conferenza stampa in cui si presentarono i dieci punti per il rilancio

così com'è ingolfa tutto e blocca la giustizia; una forte deflazione del processo civile ci darà un punto in più nella competizione e nello sviluppo. Diciamo che, rileggendo oggi quando diceva allora il ministro Tremonti, con le norme contenute nella manovra ed espunte a furor di popolo, ci siamo convinti che non solo non si riferiva propriamente a piccole e medie imprese, ma che lui era perfettamente a conoscenza di quali norme snellivano un preciso processo civile, e a quali interessi rispondevano. Abbiamo allora scorso il testo cercando di capire dove stavano i provvedimenti che spostavano il carico dalle persone alle cose. Nulla di nulla. Purtroppo abbiamo dovuto constatare che quel "prime" non stava per cornice generale, per impianto strutturale di una serie di interventi da definire magari successivamente. Quel "prime", così come tutto il provvedimento, era un semplice e demagogico artificio elettorale, nato, consumato e morto al semplice scopo di condizionare e influenzare le elezioni amministrative, successivamente perse rovinosamente da questa maggioranza. Noi non ci sottraiamo alle responsabilità che riguardano tutte le forze politiche; anzi, come qualcuno propone, noi siamo pronti a sottoscrivere un patto solenne con il Paese: definiamo i saldi, anche quelli pluriennali, e noi ci impegniamo a rispettarli, a prescindere dal ruolo che ognuno di noi rivestirà nel futuro. saldi. Lo vorrei dire a qualche collega della maggioranza che ci racconta che qualche *yacht* è sequestrato perché in qualche modo è assimilato alla normativa concernente le petroliere, non perché alcuni *yacht* dei Caraibi battono un certo tipo di bandiera, perché intestati a qualche società fasulla nata esclusivamente per questo motivo. A quei colleghi noi diciamo che il punto non riguarda i saldi, a parte la discussione sui due tempi nella politica economica. Qui il confronto doveva riguardare lo *shock* da indurre per far ripartire con nuovo passo crescita e sviluppo. In questo decreto noi, come tanti altri, eravamo incuriositi da quale sarebbe stata la frustata, la scossa da fornire all'economia italiana. Sinceramente modestissima. Faccio un esempio concreto: invece di intervenire sul turismo riportando a una funzione più significativa il ruolo del Governo nazionale e sottraendolo ai mille interessi locali, che frammentano, disperdono e annullano le potenzialità di una nostra grandiosa risorsa naturale e storica, abbiamo assistito all'indecoroso balletto sugli stabilimenti balneari. Potrei continuare così praticamente su tutti gli articoli del decreto, segnalando anche aspetti convincenti. Ad esempio, il credito d'imposta per la ricerca, che noi proponiamo con un emendamento *ad hoc* di potenziare, oppure l'adozione di un emendamento presentato alla Camera e proposto dal collega Occhiuto, del Terzo polo, in merito alla detassazione degli investimenti che si realizzeranno nel Mezzogiorno d'Italia. Tuttavia, restano una serie di questioni troppo preoccupanti. Penso, ad esempio, alle norme che riguardano Equitalia. Vedrete cosa riuscirete a scatenare voi della maggioranza con gli ennesimi tagli che riguardano il sistema degli enti locali. Per il momento, com'è possibile che non vi accorgiate che modificando in quella direzione le norme per la riscossione dei tributi comunali rischiate di mettere in ginocchio tutto il sistema dei municipi? Noi abbiamo presentato alcune proposte specifiche: la prima serve proprio ad evitare che i Comuni che abbiano affidato ad Equitalìa i servizi di riscossione si trovino nell'impossibilità di procedere alle stesse. La seconda La seconda riguarda la possibilità di sospendere per sei mesi, in particolare nel Mezzogiorno e nelle isole, e per le sole imprese in crisi, il pagamento delle cartelle di Equitalia. Abbiamo presentato poi un ordine del giorno complessivo in cui si affronta la questione della riscossione coattiva, delle vessazioni e dei tassi applicati a gente che, è bene ricordarlo, vuole pagare il dovuto e non evadere. Queste imprese, questi imprenditori, quelli che chiedono la rateizzazione delle cartelle esattoriali lo fanno perché sono in difficoltà, vogliono pagare, non sono evasori.

Noi invece come Alleanza per l'Italia abbiamo più volte presentato in questa legislatura norme per combattere la corruzione, che vanno esattamente nella direzione opposta alla vostra. È infatti nel sotto soglia che si annida spesso la corruzione e i rapporti tra pezzi di istituzione pubblica ed alcuni imprenditori più spregiudicati di altri, che in qualche modo fanno sì che il mercato resti drogato e scorrettamente operano nel settore. Praticamente qui si decide di andare dall'affidamento diretto e privato agli affidamenti ai Abbiamo poi presentato altre proposte concrete. Abbiamo individuato le risorse intervenendo sui tagli ai costi della politica. Guardate, non c'è bisogno di cedere a tentazioni demagogiche per comprendere che il Paese ha bisogno di qualche segnale concreto in questa direzione. In tale contesto, dopo che l'iniziativa del Governo non ha sostanzialmente partorito nulla sul tema dei tagli al costo della politica, noi abbiamo proposto di rafforzare la dotazione del «Fondo per il merito scolastico e universitario» e del «Fondo destinato al diritto allo studio universitario». Ci è sembrato significativo tentare di premiare il merito dei più giovani tagliando sui costi della politica e sui rimborsi elettorali. Da una parte, il Paese che studia, si sacrifica e merita, dall'altra, la cittadella della politica che fa fatica a comprendere la necessità di partecipare concretamente ai sacrifici generali richiesti a tutti. La destinazione scelta verso il merito, e in generale verso lo studio scolastico superiore e universitario, tiene conto che operiamo in un Paese dove esiste una delle più basse mobilità sociali a livello mondiale. Il figlio di operaio finisce per fare l'operaio, il figlio del professionista il professionista. Questa situazione allarma ancora di più dopo la pubblicazione degli ultimi dati ISTAT, che vedono la disoccupazione generale all'8,1 per cento e quella giovanile quasi al 30 per cento, con picchi al 46 per cento di giovani e donne del Sud. In tal senso, investire nella formazione e nel merito dei nostri giovani appare come una delle premesse necessarie per far tornare il nostro Paese a crescere: un taglio ai rimborsi elettorali dei partiti non sarebbe affatto scandaloso. Abbiamo inoltre proposto

Strano Governo, questo; strano Governo, il vostro. Viene il Presidente del Consiglio nell'Aula del Senato a chiederci di contribuire alle riforme di cui il Paese necessita e poi, alla prima occasione utile, vi presentate come al solito blindati e chiusi, quasi isolati nella vostra maggioranza. Questo provvedimento passerà il voto di fiducia e passerà anche lo scoglio del Senato:

Sud)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, seguire il lavoro parlamentare del decreto sviluppo è la storia della condizione economica e sociale dell'Italia in questo periodo così particolarmente difficile. Le misure del decreto in discussione sono volte alla salvaguardia fiscale e occupazionale delle varie aziende, con investimenti strutturali. Successivamente seguirà una risoluzione più definitiva di queste problematiche, legate anche alla forte disoccupazione, purtroppo ancora in crescita. Questi investimenti interessano soprattutto il Sud, ma voglio sottolineare che il resto dell'Italia condivide gli stessi problemi, anche se in misura minore. La situazione economico-sociale dell'intero Paese non è semplice: serve una politica volta ad eliminare gli sprechi e le inefficienze amministrative ed imprenditoriali, ma soprattutto bisogna fare tutti i tagli necessari alla spesa pubblica improduttiva. Occorre recuperare la competitività dell'intero sistema produttivo, dando elasticità al mondo del lavoro, in modo che i benefici possano emergere il più velocemente possibile. Occorre inoltre avere una grande abilità nel conquistarsi spazi nell'ambito della Comunità europea, dimostrando così la capacità del Paese di crescere in autorevolezza in originalità di esposizione ed imponendosi per la nostra qualità nella comunità stessa. È doveroso sottolineare, nel decreto sviluppo, l'interesse verso la categoria che rappresenta il nostro futuro: i giovani. Il decreto infatti contiene una serie di misure a favore della scuola, dell'università e della ricerca, attraverso le quali sarà possibile ridurre i tempi previsti per assorbire i docenti precari, risolvere il problema dell'aggiornamento delle graduatorie, sottolineo la parola "merito" - per erogare prestiti d'onore agli studenti universitari più brillanti ed istituire un credito di imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in università o enti vari. Parlando di giovani, colgo l'occasione per associarmi a quanto detto dal segretario nazionale del PdL Alfano, il quale, con molto entusiasmo, ripone la sua fiducia, come da noi sempre sostenuto nel buongoverno, sulla meritocrazia e sui giovani, considerando che sono queste le vere basi da cui il nostro Paese deve ripartire. Dobbiamo rilanciare l'iniziativa politica continuando sulla via delle riforme e dando risposte concrete ai problemi degli italiani. È bene ribadire l'importanza di valori imprescindibili quali la trasparenza, la libertà e il merito. Principi che devono tornare ad attirare l'attenzione di tutti ed in particolare dei giovani, i quali devono essere riconquistati dalla politica e per la politica. Oggi purtroppo notiamo troppo disinteresse, troppo distacco. Non è difficile capire le ragioni di questo fenomeno: i giovani d'oggi devono, infatti, scontrarsi con una realtà dominata da fattori che rendono difficili tutte le condizioni sociali. Si sentono ricordati solo durante le campagne elettorali e questo non crea in loro né stimoli né passione. Noi sappiamo invece, signora Presidente, che la politica seria, trasparente, leale, fatta da gente preparata, è il vero motore del mondo. C'è bisogno di un buongoverno perché il compito della politica è fare scelte e tra esse sono sempre da privilegiare quelle a favore delle persone che necessitano di essere ascoltate, le cosiddette classi più deboli come gli anziani, i portatori di *handicap*, i bambini. Inoltre, Inoltre, sono importanti le disposizioni del decreto in esame volte allo snellimento degli *iter* burocratici con cui spesso nel nostro Paese ci si trova a dover fare i conti. grazie all'articolo 5 sono stati dimezzati i tempi (da 60 a 30 giorni) per i controlli delle amministrazioni sugli interventi realizzati con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), che rende possibile l'avvio dei lavori nello stesso giorno in cui si presenta la domanda. È una velocizzazione rispetto alla DIA, che era la domanda di inizio lavori, la quale prevedeva invece un'attesa di 30 giorni. Al tempo stesso, però, la SCIA dà alle amministrazioni 60 giorni di tempo per verificare la presenza di tutti i requisiti, in mancanza dei quali può adottare provvedimenti di divieto di continuazione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi eventualmente già arrecati. Parlando dell'articolo 6, ossia della semplificazione amministrativa, il contenuto della norma prevede la riduzione del numero dei provvedimenti normativi, la facilitazione della comprensibilità del linguaggio amministrativo, l'accelerazione della conclusione dei procedimenti e, appunto, la velocizzazione del lavoro degli imprenditori. Si tratta di obiettivi comuni a chi come noi è fautore e promotore della semplificazione e della sburocratizzazione. La novità generale del decreto è quella di facilitare la vita delle imprese con meno adempimenti e meno ostacoli (ad esempio, il trattamento dei dati personali dei fornitori nonché i dati sensibili per dipendenti e consulenti). Nel decreto-legge in materia di misure urgenti per lo sviluppo sono previste inoltre disposizioni volte ad incoraggiare l'uso degli strumenti elettronici al fine di aumentare 1'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori come quelli di identificazione. Ciò riguarda soprattutto la carta di identità elettronica (CIE), che diventerà il documento obbligatorio di identificazione. Anche questo processo di emissione è finalizzato a semplificare l'*iter* burocratico e a ridurne i costi. Nello specifico ritengo importante sottolineare che viene soppresso il limite di età di rilascio della carta d'identità che attualmente è fissato a 15 anni. Vengono anche fissati i tempi di validità della nuova carta: tre anni per i minori di tre anni, cinque anni nella fascia di età che va dai tre ai 18 anni, dieci anni per tutti i maggiorenni. Si stabilisce inoltre l'obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori a partire dai 12 anni di età e vengono disciplinate le modalità di espatrio del minore di 14 anni munito di carta d'identità. È importante sottolineare che la CIE, la nuova carta di identità, sarà a disposizione di tutti i cittadini gratuitamente. Il miglioramento dell'*iter* burocratico riguarderà anche le strutture sanitarie dove sarà possibile pagare *on line* i *ticket* delle prestazioni sanitarie alle ASL, nella speranza che finalmente tutti li debbano pagare e non solo gli italiani. Ospedali e ASL, inoltre, potranno consegnare via *web* i referti medici. In generale ritengo opportuno sottolineare che il decreto in esame rappresenta il primo passo importante del processo d'attuazione delle misure contenute nel Documento di economia e finanza del 2011, la cui finalità consiste, da una parte , nel rafforzamento dei conti pubblici funzionale al pareggio di bilancio nel 2014 e, dall'altra, nel rilancio dello sviluppo economico. Ulteriori semplificazioni di adempimenti, di natura fiscale e non, come ho già sottolineato, vengono inoltre previste a favore sia delle imprese sia dei cittadini contribuenti. Il decreto sviluppo riguarda non solo la dimensione europea del nostro Paese, ma anche le politiche economiche rispetto ad una serie di iniziative che abbiamo avuto modo di condividere nel corso di questi tre anni come Governo e come maggioranza. Con questo decreto dimostriamo di essere coesi e determinati e di avere ben chiari gli obiettivi sui quali ci si deve muovere: l'abbattimento dei costi,

confuso e contraddittorio. Ne sa qualcosa il Governo, che, nella valutazione dell'impatto economico di questo provvedimento, ha allocato alcuni milioni di euro a copertura dell'intero provvedimento provenienti da una rivalutazione delle dichiarazioni patrimoniali dei terreni a destinazione agricola o da una rimodulazione della tassazione dei fondi immobiliari chiusi;

i nostri titoli di Stato, a nessuno di voi sarà sfuggito il fatto che il differenziale del tasso di interesse tra i titoli di Stato italiani e i *Bund* tedeschi, attestato all'inizio della crisi sui 20-30

sulle possibilità di risanamento finanziario del nostro Paese, ma anche sulle sue modeste possibilità di crescita. Il Ministro Il Ministro dell'economia ci ha detto che dobbiamo ragionare secondo logiche europee. Cerchiamo allora di declinare questa logica sull'articolato di questo provvedimento. A nessuno di voi immagino sia sfuggito il fatto che non è passato neppure un mese da quando l'Unione europea, tramite la Commissione, ha inviato al nostro Paese

questo Governo, di fronte alla raccomandazione dell'Unione europea, che invita ad adottare misure concrete entro ottobre 2011, propone una una specie di finanza elettorale. Infatti, il grosso dell'impianto che dovrà cercare di risanare realmente i conti pubblici è spostato al 2013, cioè viene lasciata questa triste eredità alla nuova legislatura, alla nuova maggioranza e al nuovo Governo. Quindi, ci rendiamo conto che anche sul piano della tenuta dei conti pubblici la maggioranza e il Governo continuano giorno dopo giorno a perdere credibilità. Un'altra raccomandazione che l'Unione europea ci ha rivolto sottolinea l'importanza di sostenere e incentivare la ricerca scientifica e l'innovazione delle imprese attraverso una estensione degli incentivi. notiamo? Questo Governo all'articolo 1 introduce il credito d'imposta per la ricerca e l'innovazione, però in via sperimentale

rispetto ai 100 milioni che erano stati promessi con la legge di stabilità. Qualcuno della maggioranza potrà dirmi che se questi milioni sono stati ridotti significa che sono stati utilizzati nel semestre precedente. Non è così, perché secondo l'articolo 1, comma 25, della legge di stabilità l'utilizzo dei 100 milioni da destinare alla ricerca e all'innovazione doveva avvenire con un decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui non c'è traccia. L'altra raccomandazione che l'Unione europea ha rivolto al nostro Paese invita ad adottare misure che aiutino a superare la segmentazione del mercato del lavoro e soprattutto a tutelare l'incentivazione dell'occupazione. Cosa fa il Governo con questo decreto? Propone il credito d'imposta per la nuova occupazione stabile nel Mezzogiorno. Dal titolo è certamente una misura importante, una misura perfettamente condivisibile; ma qual è la furbizia? Si usano delle risorse certe con coperture incerte. In un Paese come il nostro, in cui vi sono due milioni di nuovi disoccupati, un giovane su tre a livello nazionale, quattro su dieci nel Sud e una donna su due nel Meridione non trovano lavoro, trattandosi di un decreto con carattere di necessità ed urgenza, tutti quanti ci aspettavamo che il credito d'imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno avesse una attuabilità e una procedura il più possibile immediate. il Governo rinvia la possibilità di utilizzare questo credito d'imposta alle autorizzazioni e al consenso dell'Unione europea. per poter utilizzare i Fondi strutturali, i fondi FESR e i fondi FSE, si dovrà aspettare il consenso dell'Unione dell'Unione europea con tempi tecnici, con tempi burocratici e con una situazione del Paese che continua a peggiorare di giorno in giorno.

uno strumento vitale per il rilancio dell'economia turistica del nostro Paese, da Nord a Sud; tant'è che nello stesso articolo si dice anche che i distretti turistici vengono attuati

la costituzione di uno strumento importante, come poteva essere l'istituzione del distretto turistico, viene fatta nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Se andiamo a vedere nelle maglie della relazione tecnica che il Governo ha presentato, la disponibilità economica è di soli 50 milioni di euro, esattamente un sesto di ciò che il Governo ha speso per aver voluto effettuare la consultazione referendaria in data diversa da quella delle elezioni amministrative.

opere pubbliche, il Governo per la terza volta procede alla modifica del codice degli appalti pubblici e stavolta cerca di spiegarci che ciò avviene per determinare uno snellimento delle procedure, una rapidità di tempi, una riduzione dei costi, un miglioramento

Lo ha già fatto nel 2002, quando si è passati a 100.000 euro, l'ha fatto nel 2008, quando si è passati a 500.000. E non è mai successo niente!

con una differenza. Infatti, va bene la motivazione, apparentemente nobile, di voler incentivare l'edilizia, ma rispetto rispetto al piano casa precedente si va di male in peggio. Il Sottosegretario ricorderà che nel maggio 2009, in sede di Conferenza Stato-Regioni, si decise che tutto ciò che era compreso nel piano casa (l'aumento di volumetria, la delocalizzazione volumetrica delle aree, i cambi di destinazione) poteva e doveva avere un periodo limitato a soli 18 mesi, perché già da allora le Regioni paventavano il rischio che questa deregolamentazione e questa esagerata esagerata liberalizzazione delle regole potesse determinare quello che altri organismi, come ad esempio l'Istituto nazionale di urbanistica, hanno dichiarato anche in Parlamento, in audizione

una legge quadro. Questi sono soltanto alcuni degli esempi che ci spingono a considerare questo provvedimento non solo a costo zero,

che non possono più tardare. Il Paese è stanco di aspettare. Vi ha dato un messaggio forte e chiaro in occasione dell'ultima tornata elettorale e dell'ultimo

in questo decreto-legge sono presenti una serie di operazioni importanti, come l'alleggerimento della stretta sul contribuente che, in caso di cifre debitorie sotto i 2.000 euro, non vedrà più scattare le cosiddette ganasce fiscali, cioè il fermo dei beni mobili, prima di aver ricevuto due solleciti di pagamento spediti ad almeno sei mesi l'uno dall'altro. Partirà, invece, dopo 180 giorni (e non 120) dalla notifica dell'atto, l'accertamento esecutivo (misura in vigore dal 1° luglio), mentre l'ipoteca e l'esproprio della prima casa riguarderanno solamente coloro che hanno debiti superiori ai 20.000 euro, ed esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo contestata, o contestabile (comunque con obbligo per l'agente della riscossione di darne notifica preventiva). Congelato inoltre il SISTRI, il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti: per le aziende che hanno fino a 10 dipendenti, al fine di garantire un adeguato periodo transitorio,

Nel decreto non c'è il *bonus* di permanenza per gli insegnanti precari che, come Lega Nord, avevamo proposto a salvaguardia dei docenti, sia del Nord che del Sud, ai quali nel 2007 è stato chiesto di fare una scelta territoriale definitiva, che garantiva un minimo di stabilità lavorativa a loro e una pur relativa continuità didattica agli studenti. In seguito agli ultimi interventi legislativi, e in conseguenza di un'accentuata disomogeneità nei punteggi, attualmente questi docenti si ritrovano con la loro situazione rimessa in discussione. Nel decreto ci sono comunque alcune misure, da noi concordate con il ministro dell'istruzione Gelmini, e inserite nel testo originale, che vengono loro in soccorso, e la cui bontà sembra confermata dai primi dati disponibili, che segnalano un numero di spostamenti decisamente più contenuto rispetto alle previsioni. Quali sono queste misure? di cui all'articolo 9, comma 20, il quale dispone che a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, per la valutazione dei nuovi titoli conseguiti, è effettuato ogni 3 anni e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia. In precedenza, la legge n. 143 del 2004 dava la possibilità di aggiornare i punteggi e di chiedere il trasferimento in altra provincia ogni 2 anni. Si determina così un rallentamento degli spostamenti interprovinciali, e chi è in una graduatoria mantiene per almeno 3 anni la posizione occupata, senza correre il rischio di essere scavalcato da chi viene da fuori. L'articolo 9, comma 21, stabilisce inoltre che il trasferimento di coloro che vengono immessi in ruolo può essere richiesto solo dopo 5 anni di servizio effettivo e non dopo 3 anni, come consentito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 124 Con questa misura si punta contenere il fenomeno di coloro che si spostano da una provincia ad un'altra, alla semplice ricerca della nomina in relazione all'alto punteggio posseduto, attivandosi, appena centrato il risultato, per riavvicinarsi al territorio d'origine, con tutti gli scompensi immaginabili per la qualità del servizio. Pure l'assegnazione provvisoria, una volta ottenuta la nomina in ruolo, si potrà chiedere solo dopo 5 anni, a differenza di quanto previsto dall'articolo 475 del Testo unico delle leggi sulla scuola, che consentiva di presentare la domanda già dopo il primo anno di servizio, un espediente per spostarsi con facilità da una provincia all'altra, puntando ovviamente al proprio territorio. L'articolo 9, comma 17, infine, prevede «la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010-2011». L'obiettivo è l'immissione in ruolo di un contingente di docenti attingendo dalle graduatorie ad esaurimento dell'anno scolastico 2010/2011, per non aggiungere al danno della riapertura delle graduatorie anche la beffa della stabilizzazione soffiata da chi dispone di punteggi particolarmente elevati (questione tutta da approfondire, visto che in certe aree pare ne siano in possesso anche docenti relativamente giovani) a coloro ai quali lo Stato - sottolineo lo Stato - ha chiesto di fare una precisa scelta di vita impegnandosi a sviluppare la propria attività professionale in un certo territorio. Siamo relativamente soddisfatti per i posti di lavoro che con questi interventi stiamo salvando. Non è infatti rimettendo gli insegnanti delle graduatorie ad esaurimento in concorrenza tra loro che si risolvono i problemi: si toglie semplicemente il lavoro a qualcuno per assegnarlo ad altri, con tutti gli sconquassi che ne derivano. Sul *bonus*, che avrebbe garantito un buon livello di stabilità, si è scatenata l'opposizione con accuse di incostituzionalità prive di fondamento, visto che un meccanismo premiale sulla permanenza esiste già per gli insegnanti titolari, utilizzato peraltro anche da alcuni degli stessi rappresentanti dell'opposizione che accusano la nostra proposta di essere incostituzionale. Si trattava solo di estenderlo ai precari. Per essere chiari, il contratto collettivo nazionale integrativo prevede, per i trasferimenti a domanda dei docenti, un punteggio aggiuntivo come segue: 6 punti per il servizio prestato continuativamente nella stessa scuola negli ultimi tre anni; 2 punti per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio; 3 punti per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio; 10 punti *una tantum* per coloro che per un triennio (dal 2000-2001 al 2007-2008) non si sono trasferiti in altra scuola. Il *bonus* di permanenza allargato ai precari avrebbe garantito, tra l'altro, lo stesso trattamento sull'intero territorio nazionale, a differenza dei punti di Trento (su cui il TAR del Trentino ha posto il dubbio di incostituzionalità, rimettendosi alla valutazione della Consulta), che premiavano il servizio *in loco*, generando disparità di trattamento rispetto alle altre Province.

Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, quando il Governo ha annunciato il decreto sullo sviluppo

nemmeno questa volta si fa sul serio: è un provvedimento che non contiene risorse. Anzi, a dire il vero stanzia 50 milioni per

dopo tre anni di Governo nei quali abbiamo perso 4,7 punti di prodotto interno lordo,

consideriamo molto utili, tra cui mettere mezzo punto o un punto di PIL a disposizione di quei settori che possono innescare meccanismi di sviluppo in questo Paese. Guardate che è fondamentale: Paesi che sono tornati a crescere, dagli Stati Uniti alla Germania, hanno fatto così. Partiamo dai due estremi: la Grecia e la Germania.

ha iniziato ad effettuare tagli lineari, pesantissimi dal punto di vista sociale, una vera e propria macelleria sociale. Il Paese è entrato in depressione economica;

Ha varato una manovra di oltre 40 miliardi, due terzi dei quali per mettere a posto i conti, un terzo per lo sviluppo. Non è una manovra fantascientifica: due terzi e un terzo.

un po' di risorse a disposizione

perché le banche sono sempre più in difficoltà a dare finanziamenti, e che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione,

risorse nel circuito delle imprese, di quelle sane, di quelle che hanno voglia di crescere. Il Patto di stabilità.

alle liberalizzazioni sono convinto che siano a costo zero perché dalle professioni alle imprese, alle assicurazioni, alle banche siamo tornati, stiamo tornando, indietro. Ma un Paese che torna indietro nelle liberalizzazioni non è un Paese che vuole crescere.

non fa bene al Paese.

Solo questo varrebbe una manovra che si volesse fregiare del titolo di manovra per lo sviluppo. Fare un'operazione seria sul credito d'imposta per la ricerca e mettere davvero lì un po' di risorse, metterebbe in sintonia il meglio della nostra università con il meglio della nostra impresa e darebbe loro un po' di risorse a disposizione in modo da mettere in piedi progetti veri che potrebbero collocare di nuovo l'Italia all'avanguardia, come lo è stata tanti anni fa, anche dal punto di vista della reindustrializzazione (nella chimica, nella meccanica, nella energia rinnovabile). Noi abbiamo il fior fiore di imprese che se avessero un po' di risorse a disposizione per la ricerca potrebbero davvero innescare meccanismi importanti per lo sviluppo. Ho fatto un lungo elenco che sembra improponibile, ma se andiamo a fare un po' di conti, un punto o un punto

su questa strada, altro non fate che certificare la vostra distanza dal Paese. Io sono molto, molto preoccupato, perché non bisogna essere felici quando un Paese per cinque anni non cresce, ha una decrescita.

Chiudo con l'esempio della Germania: la Germania, per riuscire a fare ciò che ha realizzato, ha fatto un patto con le organizzazioni sindacali e ha fatto un Governo di solidarietà. Si sono messi a ragionare assieme. Del resto, quando si devono avviare misure strutturali e interventi di carattere strutturale - perché dopo cinque anni di decrescita decrescita ci vogliono interventi di carattere strutturale e un po' di tranquillità - bisogna ragionare assieme. Altrimenti non le fate voi le riforme, come non le abbiamo fatte noi. E probabilmente, invece, se cominciassimo a ragionare assieme, forse qualcosa di buono per questo Paese si riuscirebbe a fare.

Signora Presidente, vorrei rispondere al collega Mercatali, il quale, anche nel dibattito che avviene in Commissione

decreto-legge prevede una serie di nuove e significative misure finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell'economia. Di particolare rilievo sono le norme volte a dare nuovo impulso al taglio degli oneri burocratici attraverso la semplificazione fiscale in favore di imprese e cittadini. Credo che questa sia una volontà

la semplificazione e il rilancio delle attività imprenditoriali; interventi per il rilancio dell'edilizia privata, con il varo del nuovo piano casa; disposizioni a favore delle imprese e dei privati; norme relative al credito d'imposta per la ricerca scientifica e per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati nel Mezzogiorno; l'introduzione dei contratti di programma per la ricerca scientifica; e, infine, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, organismo indipendente a tutela dei cittadini utenti, con compiti di regolazione del mercato nel settore delle acque pubbliche e di gestione del servizio pubblico locale idrico integrato. Entrando nel merito delle disposizioni, l'articolo 1 introduce un credito d'imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università o enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento, rispetto alla media di investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Tale articolo appare di importanza fondamentale, essendo uno strumento essenziale per attivare e sostenere la competitività delle imprese italiane. In effetti, l'accesso al credito continua ad essere un ostacolo per le imprese del nostro Paese, tenuto conto della difficile congiuntura economica mondiale in cui ci troviamo. Inoltre, la ricerca diventa sempre più strategica ed essenziale. Di particolare rilevanza risulta essere l'articolo 4, che reca, tra l'altro, modifiche al codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con le finalità di ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico; semplificare le procedure di di affidamento dei relativi contratti pubblici; garantire un più efficace sistema di controllo; ridurre il contenzioso. Sono poi previste altre disposizioni molto incisive. Inoltre, le disposizioni anticipano sul piano legislativo alcune indicazioni fornite dal Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti. Tra le varie modifiche introdotte dall'articolo 4, appare fondamentale quella del comma 2, lettera *l)* che modifica il comma 7 dell'articolo 122 del codice dei contratti pubblici al fine di ridurre i tempi di realizzazione e semplificare le procedure, elevando da 500.000 a 1 milione di euro il limite di importo entro il quale è consentito affidare i lavori con la procedura negoziata a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Tale modifica appare opportuna, in quanto, pur limitando la concorrenza, determina delle ricadute occupazionali positive nelle imprese legate ai territori. È del tutto evidente che la norma deve essere gestita con senso etico e trasparenza, attraverso opportune regolamentazioni che dovranno essere adottate da ogni ente locale in modo che sia garantita l'alternanza negli inviti alle procedure negoziate. Richiamo l'attenzione, infine, sul comma 13 dell'articolo 4, che reca disposizioni volte a potenziare i controlli antimafia nei subappalti, attraverso l'istituzione, presso ogni prefettura, di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori di lavori pubblici, servizi e forniture. L'articolo 5 prevede una serie di modificazioni alla disciplina vigente, allo scopo di liberalizzare le costruzioni private, introducendo, in particolare, modifiche alle procedure delle disposizioni relative al permesso di costruire disciplinato dal testo unico dell'edilizia e alla SCIA e inoltre prevede alcune semplificazioni degli strumenti attuativi dei piani urbanistici. Nello specifico, relativamente alla SCIA e alla DIA, procedure che hanno sicuramente dato risultati positivi, si rende necessaria una ulteriore modifica per consentire una effettiva sburocratizzazione delle attività edilizie. Una delle norme più rilevanti è quella introdotta al comma 9 dell'articolo 5, che prevede che le Regioni approvino, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, proprie leggi al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio, nonché per la riqualificazione delle aree urbane degradate in cui siano presenti funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenendo conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. Tali azioni devono essere incentivate anche con interventi di ricostruzione e demolizione, che possono prevedere il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva quale elemento premiale. Tale comma crea la possibilità di accelerare l'utilizzo delle aree dismesse, che spesso costituiscono una brutta immagine del territorio, attivando in tal modo procedure veloci per il cambio di destinazione d'uso e integrando le suddette aree con il contesto urbano, rendendole omogenee. Tale procedura, inoltre, consente in tempi rapidi alle imprese che in alcuni casi rilocalizzano le attività produttive di valorizzare l'area dismessa e di reinvestire i proventi della valorizzazione dell'area nel processo produttivo dell'impresa e quindi rilanciare l'attività delle stesse. Anche l'articolo 6 prevede ulteriori riduzioni di adempimenti burocratici. In particolare, il comma 1 elenca le misure che sono disciplinate in successivi commi e ne individua la comune finalità, consistente nella riduzione degli oneri derivanti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli che gravano sulle piccole e medie imprese. L'articolo 7 specifica, al comma 1, che le norme introdotte sono volte a ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e

una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 (per gli immobili rurali ad uso abitativo) o della categoria D/10 (per gli immobili rurali ad uso strumentale all'immobile)

Le suddette norme risultano non compatibili con le norme in materia catastale e, inoltre, confliggono anche con l'interpretazione autentica introdotta dall'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207. articolo prevede infatti che le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità non si considerano fabbricati e sono dunque esenti da ICI. A tal fine, ho presentato due emendamenti soppressivi delle disposizioni suddette, emendamenti trasformati in ordini del giorno che auspico possano essere accolti dal Governo. Infine, tra le novità più apprezzabili del decreto vi è quella prevista all'articolo 9, che introduce i contratti di programma per la ricerca scientifica, con cui si intende finanziare progetti strategici di rilevante interesse per la promozione e l'attuazione di investimenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sviluppo sperimentale. L'introduzione di questa nuova forma di contratti di programma appare di vitale importanza, in quanto la ricerca tecnologica è uno strumento necessario per mantenere alto il valore dello sviluppo tecnologico in ambito mondiale. All'articolo 10, rilevante appare altresì la norma che istituisce l'Agenzia nazionale per la regolazione e creata al fine di tutelare l'interesse degli utenti, di regolare e adeguare le tariffe e di promuovere l'efficienza, l'economicità e la trasparenza nella gestione dei servizi idrici, anche in relazione alle indicazioni emerse a seguito del recente *referendum*. In conclusione, ritengo che il Governo abbia introdotto nel decreto‑legge in esame importanti e sostanziali norme, che contribuiranno ad accelerare il processo di semplificazione burocratica e ad aiutare materialmente le imprese ed i privati; esse contribuiranno sicuramente a superare la crisi che ha investito l'Europa. Infine, ricordo che le norme in esame nascono da un ampio confronto con le categorie interessate, che ne hanno sollecitato l'adozione. Va quindi un doveroso riconoscimento al Governo, che ha saputo accogliere tali istanze.

Signora Presidente, colleghi, signori rappresentanti del Governo, credo che questa lunga discussione, che si aggiunge a una riflessione abbastanza approfondita nei contenuti svolta presso le Commissioni riunite del Senato sul decreto sviluppo, sviluppo, si possa concludere sapendo che siamo in presenza di un atto che va verso la sua conclusione e che si inscrive in una e in un tentativo di governo della situazione economica del nostro Paese che non inizia oggi né finirà oggi: anzi, siamo al prologo di una manovra annunciata, che il dibattito che è stato svolto sia in Commissione che in Aula finirà per lasciare il suo esito anche al di là di questo provvedimento. Proverò a svolgere qualche riflessione. Si è detto che questo provvedimento tradirebbe il suo programma, nel senso che si tratta di un decreto sviluppo che non conterrebbe gli strumenti dello sviluppo.

di qualificazione delle procedure. Dobbiamo soprattutto essere tutti più fiduciosi sul fatto che all'interno della nostra società ci sono risorse che possono essere esse stesse motore dello sviluppo.

per fare capolino nei nostri ragionamenti. Invece, se lo Stato è il regolatore della realtà ed è la realtà che deve sprigionare le sue forze, in un concetto ben applicato di sussidiarietà, io credo che questo provvedimento (che non fa debiti), concreti. Basta leggere gli articoli per capire che non si tratta di *slogan* vuoti: dal credito di imposta per la ricerca al credito di imposta per l'occupazione dei lavoratori svantaggiati del Mezzogiorno, al tentativo di portare avanti le zone a burocrazia zero per costruire distretti di sviluppo che possano aiutare il turismo ad andare avanti, al tentativo tentativo di portare avanti una leva finanziaria nel Mezzogiorno, autorizzando quel progetto di Banca del Mezzogiorno con l'emissione di titoli di risparmio di 3 miliardi a facilitazione fiscale, alla semplificazione fiscale, burocratica e amministrativa. Certo, le riforme non si fanno per editto, lo ribadiamo; sono un processo difficile che deve rimuovere stratificazioni e comportamenti. Ma Ma escludere che in questo provvedimento ci siano fatti concreti che vanno nella direzione dello sviluppo, a mio modo di vedere, non solo è arbitrario, ma contrasta con la realtà. lo sviluppo è il tentativo della politica nel suo complesso di costruire condizioni facilitative perché le forze sane del nostro Paese si possano esprimere e la struttura burocratico-amministrativa anziché essere un freno e un impedimento diventi un fattore di potenziamento, credo provvedimento vi siano tracce interessanti. Certo, tutte le promesse possono essere tradite. Questa mattina ho fatto una verifica con il collega relatore e ho chiesto ad alcuni amministratori in materia di appalti pubblici se si erano avvalsi delle deroghe che erano state fornite in passato a proposito della soglia. Abbiamo temuto che innalzando la soglia per quanto riguarda l'affidamento dei lavori pubblici si potesse determinare uno strappo alle procedure di affidamento e quindi alla trasparenza. Ebbene, gli amministratori ci hanno risposto che

quali imprese? Come sceglierle? Per questo poi non ci sono effetti in concreto. Semmai dobbiamo capire come creare la condizione per far sì che le stazioni appaltanti polverizzate negli 8.000 Comuni italiani e nelle Province siano aiutate a svolgere i loro compiti di amministrazione: spesso è la fragilità delle stazioni appaltanti che rende deboli i procedimenti e rischia di pregiudicare anche gli obiettivi della spesa. si sottolinea la necessità di restringere le procedure e di far sì che le risorse - quelle già esistenti - si possano spendere, perché oggi il formalismo e la burocrazia fino all'esasperazione hanno preso il posto degli obiettivi (per cui anche la struttura burocratico-amministrativa più si estende sul territorio più vive una tensione e una preoccupazione, fino ad essere allarmistica); infatti, l'obiettivo della realizzazione dei programmi si perde. Il fatto che in esso ci sia un'iniezione di responsabilità io credo

formalismo e più sostanza, meno gare al ribasso che rischiano di dequalificare gli obiettivi della realizzazione delle opere; alla fine non interessa più a nessuno che l'opera si realizzi nei tempi e secondo standard di qualità. Ritengo che questo

in mille rivoli e non coglievano gli obiettivi della coesione, che pure l'Europa aveva assegnato alle Regioni dell'obiettivo 1. Io credo che tali sfide siano state obiettivamente raccolte.

La coesione è come l'amicizia: bisogna volerla entrambi per raggiungerla.

a dover fare una brutta fine in quella che era una crisi che si preannunciava estremamente pesante da sostenere per un Paese come il nostro. Invece, altre economie

tanto decantata Spagna e ad altri Paesi che si trovano in oggettive difficoltà, molto peggiori di quelle in cui versa il nostro Paese. Oggi stiamo esaminando il cosiddetto decreto sviluppo, che - l'abbiamo detto tante volte - deve fare i conti con il fatto che non può appesantire i conti pubblici che, come abbiamo detto tante volte durante questa giornata, sono avviati verso l'azzeramento del *deficit* di bilancio. Della situazione nazionale e internazionale dal punto di vista economico abbiamo già detto, e anche questo è un fattore che un provvedimento come questo deve tenere in

tenuto conto che il criterio di rotazione ha come finalità quella di evitare che la stazione appaltante possa consolidare rapporti solo con alcune imprese, mentre il principio di trasparenza comunitario richiede la predisposizione di forme di pubblicità preventiva

gli effetti distorsivi di un intervento di questo genere possano andare contro lo *slogan* che ho usato questa mattina durante la mia relazione, ossia «spendere meglio e spendere più rapidamente». Non voglio dilungarmi oltre su questo aspetto, ma ritengo che sia veramente importante sottolinearlo. L'altro aspetto, che poi è anche il secondo punto della lettera citata stamattina della presidente presidente Finocchiaro, come richiesta al Governo, era un'attenzione per quanto riguarda il ritardo nei pagamenti dei crediti delle imprese fornitrici della pubblica amministrazione. Penso che su questo siamo tutti d'accordo: l'ho già detto ieri in replica in Commissione. È ovvio, è evidente che bisogna lavorare per fare in modo che chi ha lavorato prenda i suoi soldi, perché questo è alla base di qualsiasi rapporto di tipo commerciale. Quindi, penso che stiamo parlando di qualcosa di ovvio, su cui bisogna assolutamente lavorare. Bisogna risolvere tutta una serie di problemi - lo sappiamo benissimo rispetto ai pericoli di andare contro un contenimento del debito. Rientra tutto in un meccanismo molto più ampio. Vi è anche il discorso legato al Patto di stabilità, ma anche questo è un discorso su cui si sta lavorando da tanto tempo. Sicuramente è un aspetto

perché si riesce, magari sfruttando qualche assenza all'interno della maggioranza, a contribuire a far cadere il Governo. Questo penso sia un aspetto importante che va sottolineato. Dobbiamo lavorare tutti insieme, perché il problema del ritardo dei pagamenti esiste dei pagamenti esiste e crea sicuramente delle problematiche legate anche agli investimenti stranieri nel nostro Paese. Bisogna fare in modo che si diano tempi certi, modalità certe, per cui chi ha lavorato comunque possa prendere il corrispettivo del proprio lavoro. Infine, le modifiche della riscossione dei tributi locali è l'altro tema di cui si è parlato molto in Commissione, e spesso oggi, qui in

favorire l'attività soprattutto dei Comuni medio-piccoli, tenendo appunto conto dei vincoli stringenti che hanno gli enti locali in tema di spese e di personale, che rendono difficile, se non impossibile, ai Comuni stessi assumere nuovo personale o affidare all'esterno l'attività di riscossione. Questo è un invito al Governo, che comunque è già sensibilizzato su tali problematiche, e sono certo che potrà operare nel migliore dei modi per porre

perché tutti sappiamo che, nel momento in cui mi siederò di nuovo al mio scranno, si alzerà il ministro Vito e porrà la questione di fiducia sul provvedimento.

vale a dire che con le leggi non si fa lo sviluppo. Può essere vero, credo anzi che sia vero. Temo però che con le leggi si possa fare qualcosa che disturba lo sviluppo, che è un po' invece la tradizione tipica della legislazione e anche del modo di operare dello Stato italiano. Credo che purtroppo questo provvedimento vada esattamente in tale direzione. Porto un esempio

Già nel 2008 questa maggioranza e questo Governo hanno innalzato la soglia degli appalti senza evidenza pubblica da 100.000 a 500.000 euro. Sappiamo benissimo che non c'è stata alcuna conseguenza da un punto di vista dell'accelerazione delle procedure e tanto meno della realizzazione e dell'implementazione delle opere sul territorio. Ciò che si determina con questo ulteriore innalzamento delle soglie, fino a un milione o a un milione e mezzo, sarà semplicemente un gigantesco processo di opacizzazione,

l'errore di farlo regolamentare) «i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata,» (stiamo parlando del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per chi non lo ricordasse), stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal regolamento e con la cornice programmatica definita con il Quadro strategico nazionale 2007-2013. I crediti d'imposta possono essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. Questo lo si fa (a proposito della legge che non fa lo sviluppo) con decreto non regolamentare, cioè di cui noi non sentiremo nemmeno il profumo. Allora io chiedo di avere un minimo avere un minimo di coerenza tra le parole e i fatti, perché, se volessimo dirla con una battuta, di fronte ad una cosa di questo genere, bisognerebbe evocare Totò che diceva «non esageramus». Ecco, credo che queste disposizioni davvero esagerino, perché non vanno minimamente nella nella direzione di cui avrebbe bisogno il Paese.

Credo si debba ragionare, senatore Agostini - mi rivolgo soprattutto a lei come relatore di minoranza - tenendo conto di alcuni dati, al di là delle polemiche, che fanno parte del confronto maggioranza-opposizione, che giustamente Il Governo ha dimostrato in questi tre anni di lavoro che le scelte fatte hanno sicuramente consentito al sistema Italia - non lo diciamo noi, ma gli noi, ma gli osservatori internazionali accreditati - di reggere, di essere comunque in una partita di tenuta significativa, con la possibilità, compiendo le scelte giuste, di immaginare un percorso di ripresa. ripresa. È chiaro che la sfida sta lì, e a questo mi riaggancio rispetto alla relazione di minoranza e a una serie di valutazioni che sono state rappresentate. Non siamo affatto convinti che questo confronto, così come altri che hanno preceduto il varo di questo provvedimento, non abbia maturato effetti positivi e che tutto venga travolto dall'apposizione della questione di fiducia. Non è così,

della manovra economica che è stata oggi ulteriormente presentata, con la firma del Presidente della Repubblica, al Paese. Credo pertanto che alcuni di questi temi saranno un elemento e uno stimolo utili

complicati per riuscire a determinare un risultato effettivo e virtuoso sia in termini di sviluppo che di controllo della spesa.

un elemento però è sicuramente certo: la Germania in parte cresce perché, comunque, decide di ricorrere al debito. È una condizione che noi non avremmo potuto attivare. Ad oggi la crescita del debito che è intervenuta è stata sostanzialmente determinata in parte dai tiraggi dei tassi che, ovviamente, sono, dal punto di vista della crescita, uno degli aspetti problematici che abbiamo sul nostro terreno nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Alla luce, ovviamente, di una difficoltà che altri Paesi hanno nel collocamento dei titoli, questi devono ricorrere, quindi, all'innalzamento dei tassi per renderli più interessanti. Il nostro Paese, pur godendo di una condizione diversa, come voi ben sapete, deve comunque tenere in considerazione quelli che sono flussi di carattere finanziario che condizionano questo aspetto. Altro grande elemento di condizione è la partita dello sviluppo, e su questo argomento vi sono alcuni temi che, a mio avviso, potranno essere affrontati in maniera propositiva già la settimana prossima. Uno in particolar modo riguarda la Cassa depositi e prestiti, e qui lo richiamo.

per rafforzare le politiche di intervento, e quindi la possibilità di onorare i debiti delle amministrazioni pubbliche rispetto alle imprese private, così come altre forme di sostegno al mondo delle imprese che potessero essere attivate attraverso questo strumento; ritengo sia uno degli elementi su cui potremmo lavorare nei prossimi giorni. modo, si potrà lavorare su una selezione migliore anche degli strumenti di sostegno, che vanno soprattutto nelle aree svantaggiate del Paese. Alcuni di questi strumenti sono stati codificati, e li abbiamo visti anche alla Camera; abbiamo avuto dei problemi di copertura, ma erano temi da noi già accolti e discussi proprio nell'altro ramo del Parlamento, dove vi era una condizione di agibilità, anche dal punto di vista della tempistica di conversione in legge di questo decreto, che ci ha consentito di tenere conto di queste valutazioni e dell'accelerazione degli effetti del funzionamento di questo provvedimento. Sono tutti temi che, a mio avviso, oggi trovano una significativa

Il messaggio era un messaggio che credo importante, e noi speriamo che possa essere raccolto dall'opposizione nelle prossime ore. Senatore Agostini, lei mi insegna, e d'altronde abbiamo vissuto qualche confronto qualche anno fa, per esempio sul tema del credito,

per poter trovare formule di intervento che possano essere efficaci, di orientamento efficace alle stesse realtà cui abbiamo cercato tutti insieme di garantire, in una certa fase, una fortissima autonomia, a dimostrazione del fatto che, oggettivamente,

nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei

Nella discussione sulla fiducia i Gruppi potranno intervenire per complessive 2 ore e 30 minuti, ripartite in modo non strettamente proporzionale in relazione a richieste di alcuni Gruppi di opposizione. Le dichiarazioni di voto avranno inizio alle ore 12, con ripresa televisiva diretta. Sono previsti 15 minuti per il Gruppo Misto e 10 minuti per